La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi ieri mattina, ha approvato all'unanimità modifiche ed integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 6 novembre. Questa mattina, a conclusione del dibattito sulle mozioni relative al discorso di Papa Benedetto XVI a Ratisbona, avrà inizio l'esame del decreto-legge sulla missione in Libano, che proseguirà nella seduta antimeridiana di martedì 17 ottobre fino a conclusione. Come già comunicato ai Gruppi, i tempi sono stati ripartiti. La prossima settimana, a partire da martedì pomeriggio, inizierà l'esame degli altri due decreti-legge in scadenza, in materia di intercettazioni telefoniche e di emergenza abitativa, per i quali si è ugualmente proceduto alla ripartizione dei tempi tra i Gruppi. Nella seduta antimeridiana di giovedì 19 ottobre sarà avviata, previa ripartizione dei tempi, la discussione generale congiunta dei disegni di legge relativi al rendiconto e all'assestamento del bilancio dello Stato, che proseguirà la settimana successiva. Sempre nel corso della prossima settimana sarà iscritta all'ordine del giorno la mozione Bettini ed altri sulla candidatura di Roma alle Olimpiadi 2016. Nella settimana 24-26 ottobre proseguiranno gli argomenti avviati, con precedenza ai decreti-legge. Nella seduta antimeridiana di giovedì 26 ottobre saranno incardinati il disegno di legge comunitaria 2006 ed un provvedimento per l'istituzione di una Commissione governativa di indagine sull'anziano, per il quale l'Assemblea aveva deliberato la procedura abbreviata ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento. Il calendario potrà essere integrato con documenti definiti dalla Giunta per il Regolamento, con particolare riferimento alla proposta di integrazione del Consiglio di Presidenza, e dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. Nel pomeriggio di giovedì 19 ottobre avrà luogo il *question time* sulla questione dei diritti umani in Cina. Nel presupposto dell'avvenuta votazione finale di tutti i decreti-legge nelle date di rispettiva scadenza, l'Assemblea non terrà seduta nella settimana 30 ottobre-3 novembre. Le Commissioni potranno peraltro convocarsi in relazione alle esigenze dei rispettivi programmi dei lavori. La Conferenza dei Capigruppo tornerà in ogni caso a riunirsi martedì 17 ottobre, alle ore 9, per un adeguamento di questo calendario all'andamento dei lavori, con particolare riguardo alla richiesta di istituzione di due Commissioni speciali sui diritti umani e sugli italiani all'estero e a mozioni sui flussi migratori.

Come precedentemente comunicato, a ciascun Gruppo sono attribuiti venti minuti, comprensivi di illustrazione, discussione generale e dichiarazioni di voto. Ringrazio il ministro Amato

Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi: Gerusalemme, attentato suicida, il *kamikaze* era una donna, la prima a farsi esplodere in un bar. Questo bar lo ha scelto con cura, ha fatto la propria consumazione, ha pagato il conto, si è messa vicina a una carrozzina e si è fatta esplodere. Qualche mese più tardi un pensionato sale su un pulmino di bambini ebrei e si fa scoppiare. L'anno prima, a Beslan,

Ci chiediamo: ma che Dio è questo, nel nome del quale si compiono questi atti, queste barbarie?

ci sia bisogno di guardare all'insegnamento del Pontefice, di rivedere il rapporto e il ricatto che oggi lega politica e cultura e incominciare a ragionare sui due termini opposti, quello del laicismo,

Non è possibile dialogare con il terrorismo, non è possibile dialogare con chi agisce con la forza e propugna un Dio di violenza.

a un uomo, a un progetto, ma anche al nostro modo di intendere l'uomo e l'umanità, al nostro modo di pensare all'Europa, modo di pensare all'Europa, che potremmo esplicitare con questa affermazione: «Oggi credo che questa civiltà, con tutti i suoi pericoli e le sue speranze, possa essere dominata e condotta alla sua grandezza solo se essa imparerà a riconoscere le sorgenti della sua forza, se riusciremo di nuovo a vedere quella grandezza in modo che restituisca l'orientamento e l'importanza alla possibilità di essere uomo, così minacciata, se riusciremo di nuovo a gioire del fatto di vivere in questo continente, che ha determinato le sorti del mondo, nel bene e nel male. Proprio per questo noi abbiamo il dovere costante di riscoprire la verità, la purezza, la grandezza e di determinarne il futuro, per porci quindi in maniera nuova, e magari migliore, al servizio dell'umanità». Papa Benedetto XVI, in un'intervista del 15 agosto 2005. Noi ci sentiamo di condividere quest'affermazione sull'Europa; noi pensiamo a un'Europa che con le sue radici cristiano-giudaiche abbia portato del bene all'umanità, noi siamo orgogliosi di questa Europa; siamo orgogliosi di esserne figli; siamo orgogliosi dei suoi diritti, frutto della ragione e della nostra storia; siamo orgogliosi della parità tra uomo e donna; siamo orgogliosi del diritto di poter vivere in pace; siamo orgogliosi del diritto garantito a chiunque di potersi esprimere con libertà. Difenderemo questi diritti contro il fondamentalismo islamico e li difenderemo come una nostra conquista, come il sangue dei nostri figli. Per questo riteniamo questa mozione sia un momento importante e crediamo che debba contagiare addirittura i Parlamenti europei; pensiamo anche che dobbiamo essere stanchi di di vivere il nostro essere europei come un senso di colpa, di vederci ancora come quei cattivi che hanno seminato odio in giro per il mondo o che sono la causa di tutti i mali. L'odio per gli ebrei oggi non nasce dall'Europa; oggi l'odio per gli ebrei nasce nel continente arabo. All'articolo 7 dello statuto di Hamas, trattando statuto di Hamas, trattando una dichiarazione del profeta, è scritto: «L'ultimo giorno non verrà finché tutti i musulmani non combatteranno contro gli ebrei e i musulmani non li uccideranno e fino a quando gli ebrei si nasconderanno dietro una pietra o un albero e la pietra e l'albero diranno: "O musulmano, o servo di Allah, c'è un ebreo nascosto, vieni e uccidilo"». Questo è lo Statuto di Hamas. Questo, Presidente, è lo statuto del partito a cui qualche volta molte forze del nostro Parlamento si rivolgono con fare condiscendente. Nessuno sconto a chi vuole distruggere le nostre vite, nessuno sconto a chi vuole distruggere la nostra civiltà.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'illustrare la mozione prenderò solo un minuto per consentire ai miei colleghi di intervenire; farò poi delle considerazioni in sede di dichiarazione di voto. Voglio soltanto dire che questa mozione nasce da due esigenze principali: salvaguardare la libertà religiosa e la libertà di espressione, che sono state messe a dura prova nei giorni successivi al discorso di Ratisbona;

dopo gli attacchi violenti che sono stati rivolti verso di lui in occasione del discorso che ha tenuto all'università di Regensburg. In quel discorso il Papa ha aperto con l'Islam un dialogo forte e vero, concentrato su contenuti fondamentali. Il dialogo, infatti, non può essere una parola vana, non può esaurirsi in un'affermazione generica di buona volontà. Il dialogo vero tocca i punti delicati, dove il dissenso è possibile, che devono essere affrontati con delicatezza ma anche con decisione, se si vuole cercare una comprensione più profonda ed un consenso non ambiguo. Cosa ha detto il Papa a Regensburg? Il Papa ha messo in guardia l'Occidente contro il rischio di una libertà senza verità. L'irreligione occidentale dimentica che l'uomo è fatto per la verità ed è tenuto alla ricerca della verità. La libertà, separata dalla verità, diventa mera liberazione degli istinti e delle passioni. Questo però rende, in realtà, l'uomo schiavo di se stesso. Non lo dice solo San Paolo, ma anche Aristotele: l'uomo schiavo delle proprie passioni è «servo per natura». A questa libertà senza verità, che è il punto di arrivo del nichilismo gaio dell'Occidente, l'Islam rischia di opporre una verità senza libertà, un'affermazione del potere e della centralità di Dio che non passa attraverso la libertà dell'uomo. Il Cristianesimo, che ha fin dall'inizio e nel primo movimento della sua costituzione incorporato in sé la saggezza greca, sa che la verità vuol diventare forma della vita dell'uomo per mezzo della libertà. Una verità che non fosse appropriata dalla persona umana con un atto della sua libertà diventerebbe, già solo per questo, falsa perché incapace di rendere conto della specificità dell'essere umano, che diventa se stesso per mezzo dalla sua libertà. Libertà e verità si incontrano per mezzo della ragione. Il Dio cristiano è *logos*, ragione. Il suo messaggio non sopravviene all'uomo come un comando esterno ma risponde alle attese ed alle esigenze più profonde del suo cuore. Per questo il messaggio cristiano chiede una verifica e vuol essere accolto in forza della sua intima ragionevolezza. È possibile solo all'interno del Cristianesimo questo equilibrio di verità e libertà che è l'Occidente, che è l'Europa? Può l'Islam avviarsi per il medesimo sentiero? Il Papa non nega questa possibilità. La saggezza greca muove nella direzione di quest'affermazione del ruolo della ragione anche prima e indipendentemente dal Cristianesimo. Nel faticoso lavoro di approfondimento di questa verità, che va dal prologo del Vangelo di Giovanni alla Summa Teologica di San Tommaso d'Aquino fino al documento «*Dignitatis Humanae*» del Concilio ecumenico Vaticano II, il Cristianesimo è stato in una certa fase anche aiutato da pensatori islamici. Pensiamo al valore dell'opera di Avicenna, di Al Farabi, di Averroè. Rimane tuttavia il fatto che San Tommaso ha vinto la sua battaglia all'interno del Cristianesimo, mentre Averroè ha perduto la sua all'interno dell'Islam. L'incontro dell'Islam con la modernità potrà forse avvenire se si ripartirà da questo snodo fondamentale. Questo è dialogo, dialogo vero, dialogo teologico, non parole buoniste in libertà. La proposta di un serio dialogo teologico fatta dal Santo Padre però non è stata accolta. Masse fanatizzate che non hanno letto nemmeno una parola del suo messaggio sono state scagliate contro di lui con inaccettabile violenza. Da politici dobbiamo chiederci il perché di questo fatto. La Chiesa cattolica, per l'opera di tanti sacerdoti e laici in terra islamica e per la grande testimonianza di Giovanni Paolo II, che ha difeso i diritti umani delle popolazioni musulmane dei Balcani e si è opposto ad ogni lettura dello scontro politico fra Occidente ed Iraq come crociata o guerra di religione, è il principale baluardo contro lo scontro delle civiltà. Si è voluto attaccare Benedetto XVI prima che egli possa essere conosciuto adeguatamente nel mondo islamico e prima che possa raccogliere l'eredità del prestigio del suo predecessore. L'attacco viene dall'integralismo islamico ma è riuscito a ingannare e a coinvolgere anche alcuni Governi. Proprio per questo è importante che sia forte e corale la reazione dell'Europa, della Nazione e del Parlamento italiano. In questa medesima occasione è necessario ribadire la nostra fiducia nel principio della libertà di pensiero e di parola. Condivido interamente quanto il Papa ha detto, ma ritengo che abbia diritto di parlare e di dirci altre cose, cose che gli islamici possono considerare come sgradevoli. Non è possibile rispondere a parole sbagliate, a critiche eccessive, anche alla diffamazione con la violenza, con la distruzione di vite umane, con la distruzione di chiese, rivolgendosi contro quelle comunità cristiane nei Paesi islamici che sono comunque del tutto innocenti rispetto a qualunque provocazione. Il diritto alla libertà di parola e di pensiero fa parte del processo di ricerca della verità, che è intimo al concetto occidentale di ragione. Credo che in questa occasione dobbiamo ribadire la nostra convinzione che il diritto di parola e di critica va difeso, anche se eccessivo. Certe critiche all'Islam andrebbero seppellite dal disprezzo di tutte le persone che sanno cos'è l'Islam, ma esse non possono essere fatte oggetto di minacce di morte, di violenze e di distruzioni. Credo che questa sia anche un'occasione per ribadire la nostra solidarietà alle comunità cristiane che in questo momento sono oggetto di persecuzione in tanti Paesi islamici nei quali la *Sharia* è legge. La libertà di religione è il principio della libertà umana ed è anche libertà di conversione ad un'altra religione. Non c'è Paese islamico in cui questo diritto oggi sia pienamente riconosciuto. Credo che il Parlamento italiano debba far sentire la sua voce per indicare al Governo italiano il cammino della lotta vera per la difesa dei diritti umani, che non può non implicare la difesa del diritto alla libertà di religione.

fatta dalle gerarchie cattoliche verso i credenti dell'Islam, gli Stati e le masse islamiche è avvenuto. È ripreso il grande dialogo interreligioso, lo sforzo ecumenico per il dialogo fra le culture religiose, la libertà religiosa, i diritti umani, la reciprocità della libertà religiosa. Ora sono tornate a distinguersi le voci dell'Islam moderato, dialogante (si pensi a che cosa sta avvenendo in questi giorni stessi in Marocco); sono tornate a distinguersi dagli integralismi teocratici e incominciano forse a tacere gli agitatori professionali di masse fanatizzate. Sembra essersi placato il grande incendio nato da una piccola scintilla, quella dotta citazione che, peraltro, il Pontefice già contestualizzava e già criticava, definendo troppo brusca la risposta dell'imperatore Paleologo al saggio persiano. La catechesi cattolico-cristiana sarà ora direttamente tradotta in arabo, accessibile e fruibile a chi vorrà leggere, capire, giudicare. Ma il problema ora è che cosa compete a noi, alla nostra riflessione fatta in questa sede istituzionale. Sarò brevissima, perché ho solo cinque minuti Certamente compete a noi la difesa e la solidarietà verso il Papa, la solitudine a cui è stato costretto, la campagna di diffamazione, di isolamento violenta, dolorosa. Pontefice sono contenuti molti argomenti: rapporto fede‑ragione, rapporto cristianesimo originario con l'ellenismo, evoluzione della cultura protestante; e ancor prima, potremmo dire, nel discorso di Monaco sull'illuminismo radicale, vi sono molti temi che ciascuno di noi, nella sua libertà, può laicamente condividere, rifiutare o discutere (personalmente, penso che il discorso di Monaco vada in parte rifiutato); ma la traccia che dobbiamo indicare e imprimere in questo dibattito dev'essere una traccia politica precisa, impegnativa. Se il Pontefice ha detto che la radicale estraneità della violenza ad ogni ispirazione religiosa impregnata di ragionevolezza e di umanità, perché questo è il nucleo del discorso del Pontefice (e noi sappiamo che nei secoli bui che ci stanno alla spalle la fede è stata portata con la spada, non soltanto dagli islamici), se questo oggi è il messaggio centrale, ripeto, la radicale estraneità della violenza ad ogni ispirazione religiosa impregnata di ragionevolezza e umanità, mi auguro allora che il dibattito che si svolgerà in quest'Aula oggi potenzi, per il Governo e per il mondo vasto che ci ascolta, una cifra culturale dell'Europa, un'identità europea fondata sulla distinzione laica tra Chiesa e Stato, sulla strenua difesa della libertà religiosa di tutti, sul rifiuto dello scontro di civiltà, sulla speranza che processi di democratizzazione e liberazione di grandi masse siano possibili con la sfida delle democrazie mature e sull'affermazione che non si entra nella modernità passando sotto le forche caudine delle guerre identitarie. Se l'Europa è potenza civile, noi siamo convinti che solo in questo starà la nostra speciale forza e la nostra unica autorevolezza.

Signor Presidente, signor Ministro dell'interno, mi sono posto la domanda se sia opportuno e corretto che il Parlamento di un Paese e di uno Stato laico e democratico si esprima su una questione che è e deve rimanere di dialogo tra religioni. Se invece quanto è accaduto dopo la lezione del pontefice Benedetto XVI si vuole leggere sul piano di uno scontro di civiltà, allora ritengo oggettivamente pericoloso il solo parlarne, perché ogni nostra posizione rischierebbe di essere un involontario contributo ad una logica di conflitto tra il mondo occidentale e quello islamico. Voglio cogliere comunque questa occasione per riflettere insieme a voi sulla delicatezza e gravità di un tema che costituirà nei prossimi anni la più rilevante questione riguardante la nostra convivenza. È il tema della pace che ci interpella e lo fa in un modo crudo e diretto, depurato dai folclori e dalle logiche di parte, mettendoci dinanzi al rigore della sopravvivenza e della vita, nella convinzione che ogni contrapposizione con l'Islam, ogni rifiuto di dialogo, ogni pur emotivamente comprensibile reazione ad atti contro il cristianesimo - che in una visione rozzamente sintetica viene assunto come emblema dell'Occidente - possa costituire un indiretto e magari involontario sostegno a quella parte più integralista dell'Islam, promuovendo in più l'indebolimento di tanti esponenti di quel mondo che invece credono che il dialogo fra le religioni sia il più grande segno di amore e di pace per l'umanità. Cari colleghi della minoranza, mi sono accostato a questo dibattito leggendo attentamente la vostra mozione, liberandomi da ogni spirito di parte per verificare se fosse possibile votarla - parlo della mozione che ha come primo firmatario il se essa costituisse un sostegno e un contributo alla civiltà del dialogo e della reciproca accoglienza. La questione che oggi siamo chiamati ad affrontare infatti non è se mostrare o no solidarietà al Papa cosa scontata e allo stesso tempo sentita e doverosa - né se sia giusto che il Papa possa o no esprimersi liberamente - facoltà che ovviamente è sacrosanta ma il vero nodo da sciogliere è se saremo capaci tutti, insieme, abbandonando la possibile e talvolta inconsapevole tentazione di un approccio strumentale a questa terribile questione, di trovare una strada comune, un linguaggio condiviso per affrontare un'emergenza epocale, che non svanirà tanto facilmente né tanto presto e che ci fa comprendere che il dialogo e il rispetto tra diverse culture e religioni non sono più il sogno o l'ideale di qualche intellettuale filantropo, ma una terribile necessità a cui è legata indissolubilmente la stessa possibilità di convivenza di milioni di esseri umani. Dinanzi a un terrorismo, in parte legittimato da convinzioni etiche e bene o male religiose, ogni forza è impotente; ogni arma, la più sofisticata, controproducente. La contrapposizione finisce per alimentarlo e radicarlo in strati sempre più vasti della pubblica opinione islamica. Soltanto una grande azione di cultura e di aperto, quanto profondo, dialogo potrà gradualmente fare inaridire quell'*humus*nel quale la violenza terrorista trova legittimazione. Questo non significa che si debba rinunziare ad affermare la propria cultura,

Il Papa Benedetto XVI - basta leggere il testo integrale della sua lezione presso l'Università di Regensburg - non aveva motivo per scusarsi. Eppure per ben tre volte - mai accaduto nella storia della diplomazia vaticana - è intervenuto per esprimere il proprio rammarico, dicendo testualmente: «Per

Il Pontefice sta per recarsi in Turchia non perché pensa di fare proseliti in una terra dove pure il cristianesimo delle origini ha scritto parole importanti, ma perché attribuisce a qual viaggio un'alta testimonianza della volontà e della possibilità di dialogo.

e molto recenti espresse dal Santo Padre e successive al discorso di Ratisbona : «Non agire secondo ragione è contrario alla natura di Dio». Questa è una nota che Benedetto XVI ha diffuso recentemente a commento del suo discorso, ed è chiaramente riferita all'ormai famosa frase dell'imperatore bizantino Manuele II Paleologo, che è stata determinante - lo dice il Santo Padre - in tutte le sue riflessioni e in tutta la sua vita di sacerdote e di docente. Solo ieri sera sulla pagina web del Vaticanoè stato riprodotto in maniera integrale il discorso del Santo Padre, con un'aggiunta molto preziosa ed importante di ben 13 note; 13 note di umiltà con le quali il Santo Padre ha voluto meglio spiegare anche a coloro che non hanno voluto capire - e comunque non capiranno nemmeno ora - il senso del suo discorso. Nel testo definitivo del discorso del 12 settembre vengono riprodotti alcuni sentimenti e alcune emozioni del Santo Padre. In particolare il Papa, intervenendo ormai per la quarta volta sulla questione e sulla

«Mostrami pure ciò che Maometto ha portato di nuovo» aveva detto l'Imperatore «e vi troverai soltanto delle cose cattive e disumane, come la sua direttiva di diffondere per mezzo della spada la fede che egli predicava». «Questa «Questa citazione, nel mondo musulmano», - lo ribadisce Benedetto XVI ieri sera nella sua nota - «è stata presa purtroppo come espressione della mia posizione personale, suscitando» - ecco ancora un gesto di infinita umiltà - «una comprensibile indignazione». che per noi non è comprensibile, per il Papa diventa comprensibile. «Spero» - prosegue il Papa nella notadi ieri - «che il lettore del mio testo possa capire immediatamente che questa frase non esprime la mia valutazione personale di fronte al Corano, verso il quale ho il rispetto che è dovuto al libro sacro di una grande religione. Citando il testo dell'imperatore Manuele II, intendevo unicamente evidenziare il rapporto essenziale tra fede e ragione». senza però far mia la sua polemica». Nella nota 5 il Papa illustra il brano del suo discorso, laddove dice: «L'affermazione decisiva in questa argomentazione contro la conversione mediante la violenza è: non agire seconda ragione è contrario alla natura di Dio». Dio». «Solamente per questa affermazione...» - sottolinea ancora il Santo Padre nella nota - «... ho citato il dialogo tra Manuele e il suo interlocutore persiano». Quindi, il Papa a Ratisbona, con queste citazioni, tra l'altro pronunciate nel corso di una *lectio magistralis,* e non quindi di una predica o di una omelia, voleva soltanto invitare tutti i fedeli ad avere più coraggio, ad aprirsi alla ragione: solo se ragione e fede...» - osserva ancora Papa Benedetto - «... si ritrovano unite in un modo nuovo (...) solo così diventiamo anche capaci di un vero dialogo delle culture e delle religioni, un dialogo di cui abbiamo un così urgente bisogno». Accortosi che il dialogo diventava difficile, come sappiamo, il Santo Padre ha fatto di tutto per spiegare meglio il suo pensiero all'*Angelus*, domenica 17 settembre, e in occasione dell'udienza generale del 20 settembre. Egli ha affermato che il fine ultimo era quello di evidenziare il rapporto tra fede e religione, tra ragione e fede, ribadito con accenti accorati, con il rispetto profondo per le grandi religioni, in particolare, per la religione musulmana, i cui fedeli adorano un unico dio, come i cristiani, con i quali - ha detto sempre il Santo Padre - siamo impegnati a difendere e promuovere insieme, per tutti gli uomini, la giustizia sociale, i valori morali, la pace, la libertà. Ma mentre il Santo Padre si impegnava a fornire queste spiegazioni e presentava addirittura le sue scuse - mai accaduto in passato da parte di un Pontefice - con un atteggiamento di umiltà che rasentava la mortificazione; mentre il Santo Padre andava incontro alle interpretazioni, malintese in questo modo, con profonda umiltà, dando un esempio di civiltà, suor Leonella Sgorbati veniva uccisa a Mogadiscio; minacce di morte venivano lanciate contro lo stesso Papa, il Vaticano, Roma e l'Occidente intero; devastazione a beni venivano prodotte (beni di cristiani, edifici di culto, ambasciate occidentali); mentre tutto questo accadeva, Nunzi apostolici in Paesi arabi venivano convocati per richiami per niente diplomatici; ambasciatori di Paesi arabi in Italia ed in Vaticano in particolare venivano richiamati in Patria perentoriamente.

attesa ed auspicata. Nulla è bastato perché si aspettava soltanto un'occasione, l'esca, la classica esca per farla esplodere. Il discorso del Santo Padre è stato strumentalizzato proprio in questa chiave; un discorso che purtroppo per i suoi oppositori in agguato da tempo - lo stavano aspettando - è stato un regalo fin troppo grande per un disegno - il loro - così meschino. Allora intendo concludere la intendo concludere la mie considerazioni, ricordando l'ordine del giorno G1 che il mio Gruppo ha presentato e che parte naturalmente con parole di solidarietà verso il Santo Padre, che deve essere certamente non soltanto

dichiarazioni del Presidente del Consiglio, di fronte ad evidenti contraddizioni che il Governo ha contrapposto ad un avvenimento così delicato, chiediamo di rafforzare con decisione l'azione di prevenzione e di tutela nei confronti della persona del Pontefice, che non è fatto che appartiene ad altri corpi militari vaticani, ma alla Polizia dello Stato italiano che, da sempre, si preoccupa di questo problema. Quindi, noi chiediamo che il Governo, il Ministro il Ministro competente è qui davanti a noi, metta in atto tutte le misure perché ciò avvenga nella maggior trasparenza possibile. Il secondo punto che proponiamo è di promuovere presso il Consiglio dei ministri dell'Unione Europea, presso tutti gli organismi internazionali in cui l'Italia è presente con il suo patrimonio di storia e di civiltà, il proposito di portare avanti iniziative che mirino a garantire il rispetto della libertà religiosa, soprattutto per evitare che la libera espressione della propria fede, anche in future occasioni e da parte non soltanto del Santo Padre, possa diventare motivo di discriminazione, di insicurezza e di pericolo. Parlo di professione della fede, di libertà di espressione religiosa in quanto, date le manifestazioni di inciviltà che hanno risposto al discorso del Papa, è perfino ardito immaginare che questa gente sia pronta ad accettare un principio di libertà più generale e condivisa, come

essere qui oggi a discutere di una conferenza che il Papa Benedetto XVI ha tenuto a Regensburg, l'università che lo vide docente, a conclusione poi di un ampio dibattito che ha infiammato il mondo e che ha riempito di sé pagine e pagine dei quotidiani di tutto il mondo, è la prova della persistente e forse della ritrovata rilevanza pubblica della religione e di quanto sia anacronistica una concezione della laicità che intenda rinchiudere la dimensione religiosa dell'esistenza umana nel foro interno, nella sfera privata dell'individuo. La rilevanza pubblica della religione è un dato di fatto del nostro tempo, e certamente non solo del nostro tempo, ed è ovviamente, come stiamo vedendo, un fenomeno ambiguo, tanto più quanto esso si manifesta in un contesto di globalizzazione nel quale le diverse culture vengono a contatto diretto, a confronto, a rischio di scontro. La religione può essere un formidabile fattore di scontro oppure il più potente fattore di dialogo nel mondo. È in questo contesto, complesso e per molti versi nuovo, quasi inedito, che si inserisce e nasce il pontificato di Benedetto XVI. Il dialogo religioso è per lui, per il Papa, essenziale ai fini della pace. Benedetto XVI è un costruttore di pace, nasce da qui la nostra più forte, più sincera, più sentita solidarietà contro le aggressioni che ha ricevuto. È un costruttore di pace, non un campione dell'Occidente che voglia o anche accetti il terreno dello scontro di civiltà. La croce non è un'arma e chi la usa come arma la tradisce. Basti pensare alle parole assolutamente chiare che il Papa ha pronunciato due giorni prima della conferenza di Regensburg, nella grande spianata di Monaco, quando ha concluso la sua omelia dicendo: «Il mondo ha bisogno di Dio. Noi abbiamo bisogno di Dio. Di quale Dio abbiamo bisogno? Nella prima lettura...», il Papa parla al momento dell'omelia durante la messa, «... il profeta si rivolge ad un popolo oppresso dicendo: "La vendetta di Dio verrà"». È il profeta dei cristiani, degli ebrei, non è il profeta musulmano. Il Papa continua: «Noi possiamo facilmente intuire come la gente si immaginava tale vendetta. Ma il profeta stesso rivela poi in che cosa essa consiste: nella bontà risanatrice di Dio. E la spiegazione definitiva della parola del profeta, la troviamo in Colui che è morto per noi sulla croce: in Gesù, il Figlio di Dio incarnato, che qui ci guarda così insistentemente. La sua "vendetta" è la Croce: il "no" alla violenza, "l'amore fino alla fine". È questo il Dio di cui abbiamo bisogno». Quindi, non il Dio campione dell'Occidente, che usa la spada per incrociarla contro la scimitarra, ma il Dio dell'amore, il Dio della riconciliazione. Su questo tema si è concentrata la sua lezione anche a Regensburg: il problema di come la religione abbia bisogno del filtro della ragione e di come questa abbia bisogno del lume della religione. E questo vale per il cristianesimo, come per l'Islam. Due anni e mezzo fa, nel gennaio del 2004, l'allora Cardinale Joseph Ratzinger diede luogo ad un grande dibattito con un altro grande pensatore della cultura laica tedesca, Jürgen Habermas; un dibattito che credo possa rappresentare una traccia fondamentale per la ricerca di un filo nel labirinto del rapporto tra religione e ragione nel nostro tempo. Scrisse il cardinal Ratzinger: «... mi trovo in ampio accordo con ciò che Habermas ha esposto sulla società post-secolare, riguardo la disponibilità ad apprendere e la autolimitazione da entrambe le parti», la religione e la ragione. Ci sono patologie nella religione, che sono assai pericolose e che rendono necessario considerare la luce divina della ragione come un organo di controllo, dal quale la religione deve costantemente lasciarsi chiarificare e regolamentare». La religione ha bisogno della ragione e, dall'altra parte, «esistono patologie anche nella ragione (...): una *hybris* della ragione, che non è meno pericolosa, ma a causa della sua potenziale efficacia è ancora più minacciosa: la bomba atomica, l'uomo visto come un prodotto». Aggiunge ancora: «Di conseguenza parlerei della necessità di un rapporto correlativo tra ragione e fede, ragione e religione, che sono chiamate alla reciproca chiarificazione e devono far uso l'uno dell'altra e riconoscersi reciprocamente». Questo è il grande tema del nostro tempo, attorno al quale riflette l'Occidente. Tuttavia, tale riflessione non può essere introversa, né può pensare di essere autosufficiente nella sola cultura occidentale. Scrisse ancora l'allora Cardinale Ratzinger: questa regola di base deve essere messa in pratica nel contesto interculturale della contemporaneità». Da soli non ce la facciamo, per così dire, senza il dialogo con le altre culture. È chiaro, scrisse ancora Ratzinger, che questo conflitto oggi ha per epicentro l'Occidente, ma guai se accantonassimo «le altre culture come un'entità in qualche modo trascurabile. Ciò sarebbe una *hybris* occidentale, che pagheremmo cara e in parte già paghiamo. È importante per entrambe le grandi componenti della cultura occidentale acconsentire ad un ascolto, ad un rapporto di scambio anche con queste culture. È importante accoglierle nel tentativo di una correlazione polifonica, in cui esse si aprano spontaneamente alla complementarità essenziale di ragione e fede». Questo è il senso del dialogo che vogliamo portare avanti: è un'evidente provocazione nella chiarissima distinzione dei ruoli e dei piani anche alla politica.

non è il pretesto per una rappresaglia: il pretesto dev'essere lo strumento per un allargamento della libertà religiosa in tutto il mondo, attraverso il dialogo tra le culture.

tra l'Occidente ed il mondo arabo-islamico. Guai a noi se la Turchia diventasse anziché un ponte, un cuneo all'interno dell'Europa. La Turchia deve e può diventare - su questo dobbiamo incalzarla positivamente - il ponte di dialogo. È per questo che ribadiamo la nostra solidarietà a Benedetto XVI e auguriamo a lui e a noi grandi e copiosi frutti dal suo prossimo viaggio in Turchia.

Signor Presidente, onorevoli senatori, permettetemi di dire che trovo un po' curioso questo dibattito al Senato; mi capita - pur non essendo credente - di avvertirlo, per qualche verso, anche irrispettoso. Capisco Capisco poi che c'è una strumentalità, alcune ragioni della politica che, fra l'altro, non fanno giustizia né alla storia, né alla singola vicenda di Ratisbona, ad iniziare, credo, dalle preoccupazioni che lo stesso Papa ha espresso, dalle tantissime iniziative che ha messo in campo per superare la frattura che si stava determinando - spero sia totalmente superata - con il mondo islamico. Ho letto attentamente il discorso di Ratisbona; è, a mio avviso, il discorso di un accademico, ha il limite di essere il discorso di un accademico. è quindi rischioso perché pronunciato dal capo della Chiesa Cattolica e dello Stato Vaticano. Nel suo discorso il Papa invia un messaggio al mondo moderno; dice che il mondo moderno definisce la ragione in ciò che è sperimentalmente verificabile, che è totalmente ancorato ad essa ed esclude la fede dall'ambito scientifico. Avverte una visione positivista che può creare un problema serio, tra l'altro, tra le culture, perché l'approccio razionalistico al mondo con alcune religioni crea dei problemi; essi pensano che non lasci spazio alle loro libertà religiose.

Ciò che ha scatenato la polemica, però, è l'inizio del discorso, lo citava prima il senatore Santini: la citazione del dialogo tra l'imperatore bizantino Manuele II Paleologo e un dotto persiano. Voglio citare anch'io quelle parole dell'imperatore bizantino che parla della guerra santa, la *jihad*, e dice: «Mostrami ciò che Maometto ha portato di nuovo e vi troverai solo cose cattive e disumane, come la sua direttiva di diffondere per mezzo della spada la fede che egli predicava». Mi sono stupita, onorevoli senatori, che una persona colta come Benedetto XVI incorresse in questo errore rispetto al termine *jihad*; uno dei più abusati e contemporaneamente meno conosciuti, usato solitamente per obiettivi politici e per screditare l'Islam e i musulmani. La parola *jihad* - sono convinta che voi lo sappiate, onorevoli senatori non significa guerra santa, è un termine assai complesso che riguarda lo sforzo interiore, la lotta per raggiungere un obiettivo, per farsi migliori, per bandire dalla società l'ingiustizia e l'oppressione. Quel termine viene accomunato - guardate che ciò è micidiale per un dialogo pacifico nel mondo - ai fenomeni crescenti in molte zone di guerra, alcuni terroristici, altri di legittima resistenza alle invasioni e alle occupazioni che non hanno nulla a che vedere con la guerra santa, proclamata nel 1330 da Maometto. Implicitamente il Papa ha affermato che la *jihad* è contro Dio, ha citato il giudizio durissimo e offensivo di un cristiano su Maometto, ma non ha citato la risposta dell'interlocutore, né ha fatto riferimento alla violenza delle crociate cristiane. sono esistite! Leggendo quel discorso, ho avvertito un sottile senso di superiorità della civiltà occidentale cristiana rispetto alle altre: la prima come l'unica fondata sulla ragione e alla ricerca della verità e quella musulmana in adorazione di un Dio che non ha categorie, fosse anche - cito parole del Papa - quelle della ragionevolezza. Vi sono state reazioni durissime nel mondo musulmano, dal Marocco alla Turchia, al Pakistan. Alcune sono state terribilmente offensive: caricature del Papa bruciate nelle piazze, due chiese attaccate in Cisgiordania e molte altre reazioni che non elenco perché ci vorrebbe troppo tempo. Ebbene, una come me, che pure ha una seria distanza dalle religioni e dalle posizioni di Benedetto XVI sulle donne, sulla libertà di ricerca, sulla teologia della liberazione, sull'omosessualità, ha molto apprezzato il Papa: si è mosso con generosità, senza orgogli fittizi, e si è detto rammaricato; ha attivato la diplomazia vaticana; ha divulgato una nota in cui veniva spiegato il pensiero richiamando, non a caso, la dichiarazione conciliare «*Nostra Aetate*» in cui Chiesa e musulmani vengono accomunati; ha affermato che bisogna vivere rispettando ciascuno l'identità dell'altro; ha ripetuto che la violenza religiosa va condannata da qualunque parte essa provenga o sia provenuta.

l'utilizzo di un episodio così serio per gli stessi equilibri del mondo a fini di propaganda politica sfugge francamente alla mia comprensione. L'Unione ha presentato una mozione rigorosa e rispettosa dei tanti punti di vista e dei diversi sentimenti che animano i suoi componenti. Apprezzo, in particolare, l'attenzione alle ragioni dei popoli, all'identità, al rispetto delle persone, sia per quanto riguarda le religioni che i diritti civili. Si tratta di una mozione che non è mia, ma che io riconosco: riconosco che sa parlare alle diverse sensibilità presenti. Comunque, signor presidente Marini, mi permetta di ribadire la convinzione che sarebbe stato preferibile che l'Assemblea affrontasse diversamente un dibattito così serio e delicato.

Sua Santità andava difesa dallo Stato italiano, perché in Italia c'è una maggioranza cattolica che segue il Santo Padre nei suoi ragionamenti e lo ritiene maestro di vita, oltre che maestro di vita spirituale. Detto questo, il dovere che ci compete come eletti del popolo, come Parlamento italiano, è quello di richiamarci attraverso questo episodio al rispetto della nostra Costituzione. Ricordo ai miei colleghi, e a lei, Presidente, che è di ieri la notizia di un cittadino maghrebino, il quale, portato di fronte alla giustizia italiana per delitti di una certa portata, che vanno dalle lesioni, alla resistenza a pubblico ufficiale, alla rapina, ha «I cristiani mentono sempre e io rifiuto la giustizia dello Stato italiano». Non solo - e la cosa è ancora più grave, Presidente, per chi in quest'Aula

Questo è un segnale forte e negativo che fa da eco all'altro segnale che ci viene da Milano, dove viene permessa l'apertura di una madrassa. Sappiamo cosa sono le madrasse perché conosciamo quelle del Sudan, di cui due giorni fa si è parlato, in cui bambini cristiani sudanesi vengono legati ai propri banchi per imparare a memoria l'intero Corano altrimenti non viene dato loro da mangiare.

diventato il punto principale della pastorale di Giovanni Paolo II. In quel momento già risuonavano questi primi campanelli di allarme di una forma di religiosità estrema, che neppure chiamerei religiosità ma una forma di aggressione che non tiene conto del principio secondo il quale colui che crede in Dio non può non credere in un Dio giusto e di pace, quindi non può andare a imporre i propri voleri in uno Stato altrui, non rispettando le leggi che riconosciamo nella nostra Costituzione, che giustamente abbiamo elevato ad organo di riferimento, a punto di riflessione, a punto di appoggio di tutte le leggi e di tutti i comportamenti che il cittadino, che vive e viene in Italia, deve tenere, per il rispetto di sé e del luogo che lo accoglie.

primo era quello dell'integrazione e del processo di amore e comprensione tra tutti i cristiani del mondo; l'altro era quello di una predicazione nei confronti delle altre religioni. In conclusione, Presidente, Presidente, qui non stiamo difendendo solo il Santo Padre attuale, Papa Ratzinger, ma stiamo difendendo la Costituzione italiana e i suoi princìpi.

il Papa, accusato di aver offeso l'Islam e il suo Profeta, nonostante le ingiurie e le minacce ricevute, la sua immagine bruciata in piazza, i tentativi di incendiare chiese cristiane e la concitata convocazione dei nunzi, ha offerto al mondo musulmano tre successivi attestati di stima e di rispetto, usando parole sempre più nette di chiarimento e di conciliazione. Non ha presentato scuse che non doveva, non si è difeso da colpe che non ha commesso, ha teso la mano secondo il rifiuto cristiano dell'odio e della violenza. Non so se il suo gesto alto e umile insieme riuscirà a ricomporre subito un clima di pace. La reazione degli islamici moderati ha sicuramente questo intento. Del resto, chi è convinto di avere ragione ha l'obbligo per primo di essere ragionevole. Bene ha fatto il Papa dunque a ribadire il suo rispetto nei confronti della religione musulmana; forse era stato sminuito un rischio di cui in avvenire il Vaticano dovrà tener conto. Sono tempi, infatti, in cui anche la più fortuita scintilla può fare saltare le polveriere disseminate qua e là a questo scopo. Quando Benedetto XVI, rivolgendosi stavolta all'Europa, ha ammonito che una ragione sorda di fronte al divino è incapace di inserirsi nel dialogo delle culture, aveva certo presenti le difficoltà del rapporto con l'Islam, ma non sarà questo incidente, pur clamoroso, a insidiarlo. Ed ecco il Pontefice che fin dalla sua intervista alle TV tedesche non predica, non implora, non si appella, parla sì di emergenza del male, ma anche di ragione inerte e inascoltata, condanna l'intolleranza, si interroga sui dinieghi e i divieti del cattolicesimo stesso, aprendo le porte della Chiesa a riflessioni importanti. Non possiamo non riconoscere laicamente che l'intervista di Papa Ratzinger, trasmessa il 13 agosto 2006, a veder bene intendeva dare un'idea positiva della Chiesa, nel cui ministero, cito a memoria, deve potersi vedere anzitutto l'aspetto del conciliabile e del condivisibile. Ma a noi spetta stamane di capire perché l'ormai famoso discorso del Papa ha suscitato tante e anche strumentali polemiche. Qui va ricordato che nel confronto con la pratica devozionale dell'Islam, cioè la lettura letterale del Corano, il cristianesimo offre una più lacerata e contraddittoria immagine di se stesso, favorita da una secolarizzazione che è inconciliabile agli occhi di una parte dei seguaci di Maometto, è il più grave degli scandali. Il nostro sotteso laicismo, frutto di una metodica riserva su tutto ciò che non si sottopone a verifiche di razionalità, è una storica disputa tra *fides* *et ratio*, che descrive il cristianesimo occidentale come il luogo non solo delle assimilazioni e delle compatibilità, cioè dell'incontro, ma anche della *fides infirma*, cioè incerta, insicura, messa di continuo alla prova e fonte di innumerevoli compromessi, complice - per così dire - la dimensione razionale presente anche in tanta teologia, da Anselmo e Tommaso in poi. Il *logos*, che è Dio nella folgorante apertura del vangelo di Giovanni, non è solo parola, secondo la traduzione latina di *logos* con *verbum*, è anche e soprattutto ragione. Lo ha detto con risoluta chiarezza Benedetto XVI, il Papa teologo, proprio nella sua lezione all'università di Ratisbona. Già in passato l'allora cardinale Ratzinger ricordava che il cristianesimo primitivo aveva optato per il Dio dei filosofi contro gli dei delle religioni (traggo il passo dalla sua «Introduzione al cristianesimo»). Il suo richiamo alla filosofia greca, da Platone agli stoici, per i quali Dio era il *logos*, vuole affermare che nel cristianesimo la *ratio* ha un valore più alto che in ogni altra religione: la *ratio* infatti non esclude una trascendenza anche verso il basso, verso la santa materia di Teilhard de Chardin. L'Islam invece è solo trascendenza verso l'alto, una trascendenza - intendiamoci - pura, gelosa, esclusiva. La domanda che da più parti ci si pone è se il cristianesimo, condizionato dall'avere scelto l'Occidente per la sua grande seminagione, costretto a misurarsi con la più avanzata delle scienze e a convivere con un'etica sempre più espressione culturale e sempre meno valoriale, rappresenti ancora una civiltà superiore, in grado di moderare le contraddizioni del mondo, mentre si dà spesso per scontato che l'Islam tutto quanto è un insieme di obbedienze e di intolleranze imbevute di ritualità e fanatismo, ignorando i tesori di armonia e di saggezza che la sua religione continua a riservare anche alle dimensioni civili e culturali della tradizione o via via insorgenti. Non c'è Non c'è chi non possa vedere l'abissale gratuità di un pregiudizio rimesso in vita a partire dal tragico 11 settembre, dalla barbarica strategia di una frangia fanatizzata fanatizzata e, al tempo stesso, la crociata intellettuale, politica e religiosa che da varie cattedre si è abbattuta contro l'Islam rispolverando i vecchi e logori arnesi della cosiddetta superiorità. Su queste premesse, fonti inesauribili di pregiudizi, inquietudini ed allarmi è venuto formandosi il clima che ha portato al pericoloso equivoco di Ratisbona e ai suoi non meno deplorevoli lasciti. Signor Presidente, vanno cercate qui stamattina, in quest'Aula, le ragioni che ci mettono insieme e non quelle che ci dividono. No, dunque alle estenuate e perfino pretestuose polemiche. ZAVOLI *(Ulivo)*. Un no ancora più vigoroso ai sempre in servizio appiccatori di incendi; sì, invece, al tentativo di affrontare la questione nel proposito di uscirne insieme, come mi pare possa accadere addirittura in questa stessa Aula stamattina.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, prima di qualsiasi premessa e di qualsivoglia considerazione nel merito, vorrei riprendere le parole del Santo Padre, già ricordate da altri colleghi, nella parte che tanta inutile polemica hanno suscitato. L'imperatore Manuele II si rivolge al suo interlocutore persiano semplicemente con la domanda centrale sul rapporto tra religione e violenza in genere, dicendo: «Mostrami pure ciò che Maometto ha portato di nuovo e vi troverai soltanto delle cose cattive e disumane, come la sua direttiva di diffondere per mezzo della spada la fede che egli predicava». L'imperatore spiega poi, minuziosamente, le ragioni per cui la diffusione della fede mediante la violenza è cosa irragionevole: «La violenza è in contrasto con la natura di Dio e la natura dell'anima. Dio non si compiace del sangue; non agire secondo ragione è contrario alla natura di Dio. La fede è frutto dell'anima e non del corpo». In questo punto è chiaro che il Papa vuole evidenziare l'inutilità e l'assurdità della violenza come strumento per la diffusione delle fedi religiose; vuole altresì affermare l'assoluto primato della ragione, quella che il Papa successivamente chiamerà *logos*, spiegando l'indiscusso legame tra la cultura greca e il cristianesimo. Mi chiedo, allora, che cosa ci sia stato di offensivo nelle parole del Papa: la sua accusa verso la violenza e la negazione della ragione, sia che queste provengano dal fanatismo islamico, sia che provengano da radicalismo laicista. In verità tutta la sua lezione all'Università di Ratisbona è un omaggio alla ragione, proprio perché più volte il Pontefice afferma che non agire secondo ragione è contrario alla natura di Dio. Di fronte a tutto ciò, onorevoli colleghi, appare evidente l'ignoranza, o forse anche la malafede, di chi si è scagliato contro il Papa senza aver letto, con retta intenzione, le sue parole e senza voler riconoscere il senso vero della storia. Abbiamo forse qualche difficoltà a riconoscere che l'Islam si sia diffuso con la violenza? Abbiamo forse qualche difficoltà ad ammettere che l'Islam ha cancellato fisicamente quasi tutte le stupende e storiche comunità cristiane del Nord Africa e del Medio Oriente? Abbiamo forse difficoltà ad ammettere che se i cristiani europei, a partire dal Medioevo, non si fossero opposti con forza alla violenta invasione prima araba o poi turca, oggi tutta l'Europa sarebbe ancora sotto regimi totalitari, teocratici e dittatoriali di stampo islamico? Abbiamo forse difficoltà ad ammettere che comunque nel cristianesimo, con tutti i suoi errori e degenerazioni, alla fine è sempre riuscita a prevalere la centralità della persona umana, la libertà per tutti, la democrazia e la pace? In realtà, il Papa cerca nel suo discorso tutte le ragioni del dialogo e non dello scontro; anzi, individua nel laicismo il vero e unico nemico del dialogo, perché il laicismo impone che solo la ragione positiva e le forme di filosofia da essa derivanti siano universali. Una cultura occidentale, quindi, che nega dignità alle culture religiose considerandole delle sottoculture sfida apertamente l'Islam. Il vero pericolo per i nostri vicini islamici non è certo il Papa, ma chi nega apertamente l'esistenza di Dio e si mostra intollerante verso ogni regola morale e comportamento etico. È comprensibile perciò che quasi nessuno in Europa abbia levato la propria voce insieme a quella del Santo Pontefice che - ripeto - non aveva bisogno di alcuna difesa ma di un semplice riconoscimento delle verità che da sempre proclama. Come potevano quei laicisti intolleranti, pronti a negare in ogni occasione la libertà di parola della Chiesa cattolica, pronunciarsi a favore del Papa? Non mi meraviglio di questo: è la conseguenze logica di comportamenti e mentalità ostili alla fede e, naturalmente, intolleranti. Mi meraviglio invece per il silenzio di tanti, troppi cristiani, compresi taluni esponenti politici italiani,

cercando ampie convergenze su questa materia e accogliendo un invito finale formulato dal Santo Padre al termine del suo discorso. «Il coraggio di aprirsi» - dice Benedetto XVI - «all'ampiezza della ragione, non il rifiuto della sua grandezza». È questo il programma con cui una teologia impegnata nella riflessione sulla fede biblica entra nella disputa del tempo presente. «Non agire secondo ragione è contrario alla natura di Dio», ha detto Manuele II partendo dalla sua immagine cristiana di Dio all'interlocutore persiano. È a questo *logos* e a questa vastità della ragione che invitiamo, nel dialogo delle culture, i nostri interlocutori. Ritrovare il senso Ritrovare il senso della vastità della ragione è il solo modo di far vivere l'Europa e la sua vera radice culturale, altrimenti condannata ad un arido pragmatismo o ad un assurdo fanatismo che finisce per rinunciare all'indispensabile ricerca della verità.

Ministro, onorevoli colleghe e colleghi, prendo la parola con grande difficoltà e profondo imbarazzo nei confronti del testo della stessa mozione presentata dall'Unione. Non vorrei in nessun modo provocare incidenti diplomatici o mediatici (quelli diplomatici non corrispondono alla statura della mia persona, mentre mi succede spesso di provocarne

sia - suppongo - per virtù cristiane, che per abilità di Capo di Stato, ottenendo significativi risultati in questo campo. È riuscito, infatti, ad ottenere che l'Egitto e la Repubblica islamica dell'Iran abbassassero i toni e mettessero a tacere e, in parte, sotto controllo le masse islamiche prima scatenate. Dunque, penso che nello scrivere qualsiasi documento in proposito far uso di quelle virtù repubblicane che consistono anche nell'utilizzo sobrio della ragione e delle espressioni verbali. Non appartiene ad uno stile repubblicano usare enfasi, paramenti, cerimonie. Tutto questo appartiene, secondo me, più alla tradizione delle forme assolutistiche della politica e della religione, ma questo non ci riguarda in questa sede.

avremmo dovuto intervenire nella forma che ho detto. Questo oggi mi sembra veramente eccessivo, esagerato e sbagliato, perché, tra l'altro, viene coinvolta una quantità di temi che partono dall'uso della citazione fuori contesto: basta ricordare Giansenio e Pascal per sapere che, con le citazioni fuori contesto, si può scomunicare anche la persona più pia e santa che esista. Del resto, se si volessero fare delle citazioni fuori contesto, il Deus Sabaòth, il Dio degli eserciti, è riportato nella Bibbia, non nel Corano. È stato Gesù Cristo a pronunciare la frase: «Non sono venuto a portare la pace, ma la spada».

esso se ne occupa, perché non dovrebbe, sulla base della Costituzione italiana, rilevare che in questo dialogo, benché esistano straordinarie teologhe cattoliche e protestanti (non so se ortodosse, ma è possibile) e grandi teologhe coraniche, non si vede mai un volto o una parola pronunciata da una donna in tutti i contesti in cui si riuniscono i capi delle religioni, con tutti i loro paramenti, le loro cerimonie, le loro straordinarie

tranquillo e sobrio uso della ragione. Specialmente l'Unione dovrebbe avere questa caratteristica. Se il Ministro dell'interno fosse stato ancora in Aula, gli avrei ricordato che, ad esempio, non ero d'accordo sul fatto che alle comunità islamiche italiane lui chiedesse la firma

Non si possono utilizzare due pesi e due misure. Spetta all'autorità politica agire per il rientro costituzionale delle persone che sono fuori da tali ambiti, chiedendo

oppure a chiedere che si modifichi il testo, che si trovi possibilmente qualcosa di più utile e significativo, di più rispondente ad un costume repubblicano di sobria espressione della ragione e di ricerca di quel consenso comune che è la forma laica del dialogo. A me piace che si lascino alle religioni i massimi problemi, ai quali ciascuno di noi è appassionato, e che qui vi sia più *understatement*, un

Uno dei grandi valori dell'Occidente è la libertà religiosa. Essa è una delle più grandi conquiste del Cristianesimo. La lotta dei martiri cristiani era innanzitutto una rivendicazione di libertà. Il Cristianesimo si é presentato alla storia come grande religione di libertà. Questa lotta trova il coronamento dei suoi sforzi nell'editto di Milano del 313 d. C., quando Costantino riconosce ad ognuno di professare la propria fede. La nobiltà del sacrificio dei martiri, che mai misero in discussione le leggi dell'impero e la lealtà verso l'imperatore, ma rivendicavano la libertà di credere nel proprio Dio nel rispetto e nell'amore verso coloro che credevano in altri dei o semplicemente non credevano nel Cristo come figlio di Dio, trae origine proprio dal Vangelo. Basti citare due passi fondamentali: «Rendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio» e «Se amate quelli che vi amano che merito ne avrete?». Una testimonianza altissima di questo messaggio si ritrova, per esempio, nella vita di un celebre uomo di Stato e grande santo, Tommaso Moro, che, anche quando si rifiutò di riconoscere il re come capo della Chiesa d'Inghilterra, non cessò di proclamarsi suo suddito fedele. Gli è ben chiara l'idea della libertà di coscienza che implica la libertà per ognuno di avere la propria fede, di viverla sino all'estremo del sacrificio personale, senza pretendere peraltro che lo Stato vi si conformi. La luminosità dell'esempio cristiano entra in crisi quando, per la debolezza di singole figure di uomini, si arriva ad una commistione fra religione e Stato, tra esigenze della politica e fede. Un passaggio chiave sta nella dichiarazione di Teodosio I che proclama il cristianesimo religione ufficiale dell'impero, ma già prima lo stesso Costantino aveva dato avvio alla pericolosa prassi di convocare e presiedere lui stesso i concili dei vescovi perché giudicava interesse dello Stato controllare la religione. É il cosiddetto cesaropapismo che avrà poi nel medioevo l'altra faccia della medaglia, allorché Papi e vescovi diventeranno pure loro autorità politiche secondo una prassi già inaugurata proprio nell'ultimo periodo dell'impero romano, quando ai vescovi erano state affidate funzioni giudicanti nei processi comuni. Si dovrà aspettare Locke e i suoi fondamentali saggi sulla tolleranza e sull'intelletto umano, oltreché l'orgogliosa rivendicazione dei Padri pellegrini culminata nella rivoluzione americana per ritrovare lo spirito originario della società cristiana e riaffermare la libertà religiosa di ogni fede davanti allo Stato. La libertà religiosa è il pilastro della dottrina della Chiesa. Ricordiamo, per esempio, la celebre affermazione di Giovanni Paolo II quando ebbe a dire che la libertà religiosa è la base di tutte le libertà. Tutto questo percorso è mancato all'Islam. Vi è di più. Il Corano è piuttosto un libro di fede e insieme un grande trattato giuridico che intende dettare regole e sanzioni da applicarsi all'interno della società a tutti indistintamente. Da qui l'idea che domina fra i credenti musulmani che la *Sharia* debba essere legge civile. Da qui trae origine anche la totale commistione tra fede e politica, fra Stato e religione nei Paesi islamici, da qui la difficoltà ad accettare il pluralismo religioso. Una riflessione e un'interpretazione del Corano all'insegna dell'accettazione della libertà religiosa e della separazione tra Dio e Cesare sono tuttavia il presupposto fondamentale perché si possa arrivare stabilmente a una pacifica convivenza e ad una feconda integrazione tra islamici e non nelle società occidentali. Alla base di questa accettazione vi è il ricorso alla ragione, richiamato proprio dal Papa a Ratisbona. Il problema è che l'Islam non ha un Papa, vale a dire un unico capo capace, con la sua riconosciuta autorità, di fondare definitivamente una certa lettura dei testi sacri. Probabilmente solo la fermezza e l'unità di coloro che credono nella libertà e nell'integrazione, nel pretendere una diversa capacità di ascolto e d'accettazione della diversità dei giudizi e nel contempo

Questo è il punto. Non possiamo dividerci; non possiamo tacere ogni qual volta sia minacciata la libertà religiosa che significa il diritto di esprimere la propria fede, di darne testimonianza, di sostenere con argomentazioni e senza violenza la verità del proprio credo religioso e la sua differenza rispetto a quello altrui. libertà religiosa è libertà di professare e va di pari passo con un'altra libertà fondamentale: la libertà dalla paura, dall'intimidazione, dalla minaccia e dalla sottomissione. É in nome di questi ideali di libertà che ora chiediamo un impegno del nostro Governo a farsi interprete di un'istanza che corrisponde ai valori più profondi della nostra Costituzione, della nostra storia, della nostra stessa identità e che presuppone ovviamente, da parte di chi ci governa, un'adeguata consapevolezza e condivisione di quei valori e dei rischi a cui essi sono sempre più esposti

«datemi lo scritto di chiunque e vi assicuro che isolando una frase dal contesto sarò in grado di inviarlo al Patibolo». Queste erano le parole di Joseph Fouchè, ministro della polizia sotto Napoleone. Ed è quello che è accaduto poche settimane fa. Infatti, mentre da noi non si riuscivano a placare le polemiche, sono bastati due giorni al presidente dell'Iran Mahmoud Ahmadinejad per assumere una nuova posizione che esprimeva rispetto per il Papa, suggerendo lui che le parole di Sua Santità fossero state riportate da molti in maniera scorretta. Non potremo facilmente tornare indietro, comunque, rispetto alle grandi parole pronunciate dal Pontefice in terra di Germania, certamente non per l'umiliante polemica che ne è seguita, alimentata ad arte dai *media* occidentali, ma per la sfida che il Papa ha lanciato alla modernità e riguardo all'uso e alla concezione della ragione. Il Papa non è andato in Germania per una missione diplomatica in cui ogni singola parola è resa asettica dalle esigenze di adeguarsi alle regole oggi imperanti della politica corretta. Ogni sua tappa è stato un pellegrinaggio alle sorgenti della fede. Quando ha parlato a Ratisbona era pienamente consapevole di non parlare in un *talk* *show* ma stava svolgendo una *lectio magistralis* e l'ha affrontata sapendo di parlare a saggi sul tema delicatissimo del rapporto tra fede e ragione e, in un certo senso - ripeto - in un certo senso, ha posto sullo stesso piano Islam e Occidente, affermando che il rapporto tra fede e ragione è entrato in crisi per entrambi nel momento in cui ci si è distaccati da quel tramite straordinario, la filosofia greca, che meglio di qualsiasi altra esperienza aveva proprio avvicinato e fatto dialogare questi due elementi. È importante allora riannodare questo rapporto strappato tra fede e ragione perché se la ragione si separa da Dio perde la sua naturale tensione all'infinito e se la fede rinuncia alla ragione o si affida ad un Dio irragionevole genera violenza.

che attacca a testa bassa tutto ciò che, anche da lontano, richiami alle certezze di una parola che forse qui non è ritenuta politicamente corretta ma che oggi voglio usare, cioè la verità. Non l'incontrovertibile realtà dei fatti, perché quella è la realtà, ma l'incontrovertibile realtà dei valori che si fondano sul diritto naturale. E quando parlo di verità so di non offendere la sensibilità e la laicità di tanti colleghi non credenti, che però non rifiutano la realtà del diritto naturale, sia pure a cielo chiuso, cioè senza Dio, perché ben sanno che parlo di verità costantemente illuminata da tutti i passaggi della ragione. So invece di offendere l'ottusità laicista di un relativismo etico a tutti i costi, che ci impone di considerare tutto uguale al contrario di tutto. E se anche qui riecheggia, più o meno velatamente, uno scontro di civiltà che certamente non abbiamo voluto noi, di certo l'incontro è tra persone; le identità sono importanti,

allora difendiamo il diritto di parola del Papa perché è anche il nostro diritto e permettetemi di concludere con le parole riportate dal Papa in un breve discorso di Manuele II partendo dalla sua immagine cristiana di Dio all'interlocutore persiano, sostenendo che "non agire secondo ragione *(*con il *logos)* è contrario alla natura di Dio". È a questo grande *logos*, a questa vastità della ragione, che invitiamo nel dialogo delle culture i nostri interlocutori. Ritrovarla noi stessi, sempre di nuovo, è il grande compito e la grande sfida dell'umanità. *(Applausi

La *lectio magistralis* di Benedetto XVI all'Università di Ratisbona, dove era stato docente per molti anni e in cui ritornava nelle vesti di Pontefice, ha avuto un uditorio davvero universale. Le sue parole pronunciate in un luogo e in un tempo ben precisi, davanti ad un uditorio che aveva caratteristiche ben definite, hanno acquistato in tempo reale una risonanza senza limiti né di spazio né di lingua. Tutti abbiamo potuto leggerle e ascoltarle allora e molti di noi nell'arco delle settimane successive abbiamo voluto rileggerle e ragionarci su con serenità, cercando di penetrarne il senso. Al di là dell'impatto mediatico iniziale che ha creato intorno a quella lezione un chiasso assordante, emotivamente carico di reazioni assai diverse, siamo stati sorpresi dall'intensità con cui il mondo intero ha preso posizione, confermando l'interesse generale con cui viene accolto il Magistero della Chiesa, soprattutto quando parla attraverso il Santo Padre. La maggior parte delle persone, cattoliche e non cattoliche, colte e meno colte, praticanti e non praticanti, si sono schierate accanto a Benedetto XVI, ne hanno preso istintivamente le difese identificando immediatamente il senso di quella frase in cui fede e ragione erano chiamate in causa per aiutare a comprendere meglio il valore della religione, di ogni religione, e l'impegno che richiedono ad ogni uomo che cerca rettamente Dio. Ad alcuni invece, come è noto, la stessa citazione contenuta nella frase incriminata è sembrata svalutativa, per cui si sono schierati dalla parte di un Islam violento e aggressivo, che ritenendosi offeso dalle parole del Papa, ha minacciato pesanti atti di rivalsa e ne ha preteso le scuse pubbliche, anch'esse globali. Sappiamo tutti con quanta delicatezza, ma anche con quanta tempestività e con che assoluta chiarezza il Santo Padre ha voluto spiegarsi e spiegare il senso di quella citazione, offrendo a tutti noi una ulteriore opportunità per cogliere appieno il suo pensiero. Il Cardinal Poupard, presidente del Consiglio per il dialogo interreligioso, ha definito quel testo come: «una mano tesa, perché rivendica il valore delle culture religiose dell'umanità, tra cui l'Islam...». Il punto centrale della lezione è stato il rapporto tra fede e ragione, nella consapevolezza che nessuna possa prescindere dall'altra, ma che ognuna debba occupare il posto che le è proprio. Ratzinger infatti nella sua lezione ha detto con chiarezza: «Una ragione che di fronte al divino è sorda e respinge la religione nell'ambito delle sottoculture è incapace di inserirsi nel dialogo delle culture». Benedetto XVI ha voluto ancorare ad un retto uso della ragione ogni possibilità di dialogo, indispensabile per confrontarci con la complessità della cultura contemporanea, con le sue contraddizioni, a volte solo apparenti, ma indispensabile soprattutto quando tra gli uomini, a volte anche tra di noi, le diversità sembrano rappresentare una barriera e non più una risorsa. Cercare con pazienza il punto di incontro, parlare con chiarezza, cercare di spiegarsi senza timori e senza pregiudizi, ascoltare con attenzione e con rispetto un punto di vista diverso dal proprio o da quello del proprio gruppo, progettare soluzioni il più possibile condivisibili, è un esercizio che dovrebbe dare alla politica un suo alto valore di servizio. L'intelligenza umana è fatta per questo: per interrogarsi sui problemi della quotidianità e su quelli che assumono rilevanza esistenziale, come sono ad esempio quelli che hanno per oggetto il rapporto dell'uomo con Dio e con gli altri. Per questo, mentre esprimo a nome di moltissimi dei presenti che non sono potuti intervenire nel dibattito la piena solidarietà a Benedetto XVI, voglio anche ringraziarlo per la sua incessante catechesi che ci avvicina alle verità di fede e ce ne svela il senso, mentre ci mette davanti alle nostre responsabilità anche sotto il profilo politico, prima tra tutte quella di garantire ad ognuno piena libertà religiosa. Per questo, e mi avvio a concludere, ancora una volta, dico grazie al Santo Padre, e aggiungo che a molti di noi piacerebbe ascoltarlo e ricevere direttamente da lui una lezione sul rapporto tra vita di fede e vita politica, tra laicità e religione. Chissà che questa non possa essere un'opportunità per chiedergli di ricevere quanti di noi lo desiderano davvero!

credo che tutti i colleghi abbiano ascoltato con molta attenzione la discussione delle diverse mozioni e del dibattito; io comunque l'ho fatto e mi rendo conto in particolare di due cose, e per questo chiedo una breve sospensione. Vi è molta più convergenza istituzionale di quanta probabilmente non fosse ipotizzabile all'inizio del dibattito

Vi è un senso di libertà religiosa che rappresenta il motivo comune della nostra appartenenza, anche della nostra diversa idea sulla religiosità e, ovviamente, in questa comune idea della libertà di religione esiste una specificità della religione cattolica, in base agli articoli 7 e 8 della Costituzione. Quindi, mi sembra opportuno che il voto finale se, come mi auguro, sarà unanime, possa contemporaneamente essere un voto dal quale nessuno

Signor Presidente, onorevoli senatori, ho ascoltato con grande interesse il dibattito che si è svolto sinora.

davanti ad un tema così difficile e delicato come questo (tanto difficile e delicato da farmi dubitare, a volte, della della pertinenza di questa sede, il Senato della Repubblica, nel valutare dall'interno le parole del discorso di un Pontefice), che cosa sarebbe successo se al termine del dibattito mi fosse stato chiesto quale mozione il Governo preferiva su questo argomento.

e che su questioni come queste vi sia una convergenza di sentimenti e di posizioni che vedo, fortunatamente e utilmente, essersi realizzata nell'approntamento di un ordine del giorno che possa essere approvato da tutti.

per il nostro futuro, per la nostra stessa civiltà, per il rapporto di questa civiltà con altri; vanno al limite e al di là di quello che ciascuna delle nostre istituzioni può fare da sola.

su questo tema ciascuno di noi impegni se stesso; il Governo, naturalmente, per la sua parte. È evidente che siamo alle prese con un tema che va al di là del dato meramente istituzionale: il rapporto fra culture e civiltà, la libertà di religione, la libertà di ciascuno di esprimere la propria fede religiosa, le differenze che tuttora esistono tra quello che chiamiamo Occidente e quello che viene chiamato Oriente, il rapporto fra fede e ragione, il rapporto tra fede e fanatismo. Tutti temi su cui, se troppo possono i Governi, vuol dire che sono mal risolti e mal affrontati. É bene, quindi, discuterne in modo aperto;

ricevere da Governi di altri Paesi la richiesta di chiedere delle scuse per ciò che aveva detto il Santo Padre, percepire il bisogno che tali scuse fossero espresse in ragione non di una profonda convinzione religiosa, ma - lo dico senza peli sulla lingua - in ragione della paura: non eccitare una tigre che può portare ad atti di terrorismo nei nostri confronti, non eccitare, nei Paesi i cui Governi richiedevano di chiedere delle movimenti che possono costare a quei Governi il posto alle elezioni successive. Allora, che facciamo? Chiediamo scusa, i moti si placano e diciamo che questo è dialogo tra le civiltà e dialogo tra le religioni? Non è dialogo tra le civiltà e dialogo tra le religioni; è espressione di parole caute dettate dalla paura, parole caute dettate dalla paura, che però non sono dialogo e non debbono sostituire il dialogo, debbono essere superate da qualcosa che permetta un giorno al mondo di superare questa assurda situazione nella quale vi sono moti violenti e si mettono a repentaglio vite umane in ragione di cose che vengono dette e che attengono, sia pure, alla materia religiosa. Accetto che vi siano sentimenti religiosi che si esprimono decisamente in culture diverse. Noi siamo abituati a un Dio che, evidentemente, non si offende se ogni tanto lo facciamo apparire in qualche vignetta.

religioni?». L'ho trovata pertinente perché, in qualche modo, inventando le religioni Dio ha inventato una capacità di lite tra gli esseri umani che probabilmente non era nelle sue intenzioni. Capisco che altri possano ritenere questo un modo irriverente di trattare la divinità. Non comprendo, tuttavia, e non posso accettare che, in ragione di tale irriverenza, possano scatenarsi dei moti violenti che addirittura mettono a repentaglio la vita di chi la pensa diversamente e accetta tutto questo. Allora, sono pronto a dire, come altri hanno detto nel nostro e in altri Paesi europei, che non dobbiamo limitarci a chiedere scusa per sedare i tumulti momentaneamente.

su come dobbiamo impostare il rapporto con chi la pensa diversamente da noi per evitare che ciò accada in futuro, per far in modo che ragione accompagni sempre le manifestazioni di fede. È evidente che che dobbiamo renderci conto e prendere atto di qualcosa che ci riguarda profondamente e cioè del rapporto che storicamente c'è stato tra noi e altri che oggi ci vedono in un certo modo. modo. Se c'è una cosa che dobbiamo fare, è saper storicizzare noi stessi, rendendoci conto che la contemporaneità ha fatto convivere, l'uno a fianco dell'altro, nello stesso tempo, Paesi, culture, civiltà che in realtà vivono tempi diversi. In chi vive fuori del cosiddetto Occidente vi è ancora l'immagine dell'Occidente che è stato, non di quello che noi giustamente pensiamo di essere. un filone di studi, tanto occidentali quanto orientali, che si autodefinisce «studi *post* coloniali», che mette bene in evidenza le radici di quel sentimento di umiliazione che si prova spesso in Paesi nei quali noi siamo stati poteri coloniali davanti a ciò che noi, ancora oggi, siamo e facciamo e la percezione di ciò che noi siamo e facciamo come modi per affermare una nostra superiorità. Ho parlato non con politici, ma con filosofi del mondo arabo che considero moderati, i quali sono tuttora pronti a identificare nostre posizioni dottrinali (non politiche) come espressione di un modo, per noi, di affermare la nostra superiorità. Il che genera un sentimento di costante frustrazione nei nostri confronti che proietta su di noi un'immagine negativa figlia di un'immagine passata. L'idea dell'Occidente come male e corruzione, che ha tante pezze d'appoggio in taluni modi di vita della nostra civiltà occidentale, è largamente figlia dell'immagine della città in cui si insediava il potere coloniale e della corruzione, prostituzione, pessimo uso del danaro che in questa città coloro che vi vivevano prima vedevano come portato dai colonialisti occidentali. Leggete quanto un grande autore moderato qual è Avishai Margalit sulla città corrotta e vedrete che buona parte di quello che il mondo islamico attribuisce a noi, in termini di corruzione dei costumi e della vita, è figlio della visione della città in cui si era insediato il potere coloniale. C'è un' arretratezza di costumi con la quale dobbiamo fare i conti? So bene, come è stato detto dal collega che ha parlato per primo a nome della Lega, noi ai tempi della Resistenza non facevamo cose che vengono fatte oggi, ma tre o quattro secoli fa le facevamo, anche se da noi non c'è mai stato il fenomeno terrificante del kamikaze che uccide sé stesso per uccidere altri.

Buona parte del mondo islamico vive oggi una fase di arretratezza storica, ma anche di dogmatismo oscurantista nel leggere la propria religione,

che era probabilmente alle origini del *logos* che stava in principio, dopo secoli nei quali l'abbiamo storicamente negato. negato. L'odio verso gli ebrei che si legge nei libri di Hamas è un odio che la cristianità ha malamente alimentato, violando i princìpi fondamentali del suo Vangelo, contro gli ebrei vittime dei *pogrom* in tanti dei nostri Paesi, nei secoli passati. Di ciò dobbiamo essere consapevoli; dobbiamo sapere che nella storia i messaggi religiosi sono stati affidati a uomini di poca o di pessima fede, che ne hanno fatto uso per brandire la religione in nome dell'odio, e non in quello dell'amore. Noi condanniamo la *Jihad*. Noi oggi affermiamo che la guerra santa non è ammissibile e molti di noi sostengono che la guerra non è mai ammissibile, santa o non santa che sia. Tuttavia, in nome della cristianità sono state fatte le guerre sante sono stati benedetti labari, truppe e quant'altro. Noi abbiamo il beneficio storico di averlo superato, ma altri non lo hanno ancora fatto. Se ci manca questa consapevolezza, se ci manca la capacità di chiedere scusa non per un discorso di Regensburg, ma per il nostro passato; se ci manca il coraggio che ebbe sua santità Giovanni Paolo II, andando davanti a quel Muro a chiedere scusa per gli errori passati, sarà difficile

infatti, che spesso nei nostri Paesi si rischia di creare un conflitto manicheo tra due errori: quello di brandire la nostra religione contro altri e quello di ritenere che tutto, in nome della correttezza politica, sia ammissibile in quanto proviene da altri, e che quindi tutto dobbiamo accettare come espressione di un'altra civiltà. Questi due errori sono simmetrici. Noi abbiamo il diritto-dovere di reagire contro la violenza in nome di una qualunque religione. Non dobbiamo ritenere che quella violenza sia espressione di una civiltà che abbiamo il dovere di rispettare. Allo stesso tempo, dobbiamo evitare di attribuirci una superiorità precostituita, quasi che fossimo, o fossimo sempre stati, immuni da errori. Se saremo in grado di riconoscere che, nella sua storicità, qualunque religione, compresa la nostra, può essere stata tradita, saremo meglio in grado di capire che anche l'Islam viene tradito e saremo meglio in grado di cooperare con coloro che nel mondo islamico lo considerano tradito. Se c'è una cosa che trovo culturalmente inammissibile, oltre che politicamente nefasta, è la domanda frequente: dov'è l'Islam moderato? Ecco, l'Islam moderato, tanto per cominciare, lo abbiamo in casa. Lo si ritrova nelle migliaia e migliaia di donne che sono venute come immigrate in Italia, che non sono ancora cittadine italiane e che sono quindi tuttora soggette alle leggi del loro Paese, che desiderano ardentemente poter essere come noi, che desiderano ardentemente non essere assoggettate ad una potestà maritale arbitraria, che desiderano poter non essere segregate in casa, dove spesso i loro mariti finiscono per rinchiuderle. Loro sono islamiche e sono orgogliose di esserlo; considerano il loro essere islamiche più che compatibile con l'affermazione dei diritti della persona e della donna e più che compatibile con la negazione dell'uso violento del potere maschile più casi, con l'uso violento della religione. Mi sono battuto in silenzio insieme a molti altri per un amico, un intellettuale iraniano,

questo professore è nuovamente libero e può continuare insieme ad altri a lavorare per un dialogo tra le civiltà.

Dobbiamo fare in modo che in quel mondo chi eccita alla violenza venga progressivamente messo nella condizione di risultare minoritario e isolato. Questo è il mondo del quale abbiamo bisogno,

compito ritornare ad una lettura dei testi religiosi che sia tale da farne - come possono essere - il fondamento della pace.

A volte leggo troppo odio nel modo in cui si leva la voce nel nome della cristianità e sento in ciò il tradimento di quel messaggio che oggi - l'ho sostenuto - dà alla cristianità una posizione preminente nel mondo, proprio perché fede e ragione hanno trovato in essa una capacità di connettersi che storicamente e non in linea di principio altri hanno incontrato o stanno incontrando difficoltà a stabilire allo stesso modo e nella stessa misura. Ciò è avvenuto perché la cristianità ha appunto in in questo senso dell'amore per l'altro e del riconoscimento dell'altro, quale che sia la condizione in cui l'altro si trova, la sua caratterizzazione fondamentale. Per questo va difeso il Papa; per questo bisogna non chiedere scusa per ciò che ha detto; ma per questo bisogna non rompere, bensì costruire legami con chi possa non condividere la verità del Papa, ma condividere il senso di dialogo, e quindi di pace, che quello porta con sé. Non arriveremo mai, in un mondo con più religioni, ad avere delle verità religiose condivise (questo mi sembra assolutamente ovvio), ma possiamo fare in modo che le religioni (ciascuna con la propria verità) concorrano ad un tessuto di pace e di riconoscimento reciproco. Detto questo, mi limito ad aggiungere che il viaggio di Sua Santità sarà seguito da noi con la massima attenzione. Già oggi seguiamo con particolare attenzione - in questo caso parlo non a nome del Governo in generale, ma in particolare del Ministero dell'interno ciò che accade lì intorno. In ogni caso quelle parole sono state pronunciate, quella citazione è stata fatta, quel tipo di reazione è intervenuta e può essere il serbatoio di quello che in gergo è definito attentato vendicativo. E noi, consapevoli di questo, pur non avendo, ve lo posso assicurare, nessun segnale specifico in questo momento, stiamo molto attenti a che nulla possa accadere. Non possiamo seguirlo in Turchia. Qui non siamo competenti. È affidata principalmente alla polizia turca e allo stesso Vaticano la definizione dei termini che possono garantire la sicurezza di Sua Santità in quel viaggio, ma sono contento che lo faccia e penso che la sua scelta di mantenerlo in un Paese che si trova ai confini dell'Europa, ma che è anche quello di San Paolo, significhi qualcosa non so se per il futuro dell'Europa - me lo auguro - ma di sicuro per quello del dialogo tra le religioni. In questo senso, signor Presidente, con

ci troviamo di fronte ad un ordine del giorno «plurimodificato». L'ultima modifica è quella che trasforma il Santo Padre in Pontefice,

con quello di «Pontefice», sottolineando che il ministro Amato, nel suo discorso, ha continuato a chiamare il Papa «Sua Santità». Si tratta, quindi, di un atto di solerzia che non condivido e non capisco. Posso immaginare - come ci insegna il collega che sta normalmente seduto qui in basso - che pensando male ci si indovina sempre e che dunque l'iniziativa sia partita dalla parte opposta di questo schieramento. Allora, ho pensato male e chiedo scusa, però vorrei chiedere a chi ha assunto tale iniziativa di rendersi interprete e promotore di analoga iniziativa al fine di chiamare il Dalai Lama con un appellativo differente da «Sua Santità»,

Presidente, ovviamente è una questione delicata, ma voglio dire al collega che mi ha preceduto che questa iniziativa è venuta personalmente da me per una ragione di ordine strettamente costituzionale:

Signor Presidente, l'equivoco circa la sostituzione dell'espressione «Santo Padre» con l'espressione «Pontefice» e il fatto che per sbaglio la copia consegnata alla Presidenza non contenga la sostituzione della parola «Santo Padre» con «Pontefice» è addebitabile a me. Ho sbagliato io. Non so se cogliete il fatto che da questi due equivoci forse quello che emerge con grande evidenza è l'assoluta solidarietà di tutte le forze politiche rappresentate in questo ramo del Parlamento su quell'ordine del giorno.

che è sparito il termine «integralismo», come se non appartenesse al vocabolario della lingua italiana, sostituito dall'altro questo non voglia dire che l'integralismo sia tollerato dall'Assemblea. Vorrei che questo fosse esplicito e che tutti sapessero che gran parte

quindi non da un senatore di sinistra. Io personalmente ritengo che l'integralismo sia un insieme, un complesso di filosofia e di pensieri che, di per sé, avversiamo, ma evidentemente non tutti ritengono questo. Rispetto le altre opinioni. Il senatore Pirovano non si preoccupi se abbiamo lavorato con grande capacità di ascolto reciproco e di confronto reciproco. Formalmente questo ordine del giorno porta la firma di tutti i Capigruppo e allora sono loro che, nel loro giudizio, tengono in piedi questo strumento nell'Aula. Mi pare che non ci siano obiezioni tra i Capigruppo; non ci sono obiezioni nemmeno al fatto di usare, per la motivazione molto laica sottolineata dal senatore D'Onofrio, la parola «Pontefice». Se è così io credo che, con il consenso dei Capigruppo, possiamo procedere

È chiaro: su problemi della portata di quelli di cui stiamo discutendo, come la linea da seguire nella lotta contro il fanatismo islamico, contro la *Jihad,* la necessità di tenere aperto il dialogo, esiste nelle diverse forze politiche presenti nell'Aula una varietà di posizioni e di sfumature anche importanti, all'interno - credo - di una convergenza sostanziale. In questo momento ci troviamo alla vigilia del viaggio di Benedetto XVI in Turchia e credo che la sostanza, a cui vorrei richiamare tutti, sia che il Parlamento italiano, il popolo italiano, unanimemente sostengono lo sforzo di pace del Papa, difendono il suo diritto a parlare della verità, riconoscono l'importanza che la sua azione, e questo viaggio in modo particolare, hanno per instaurare un clima di libertà nel mondo, manifestano solidarietà ai cristiani perseguitati, richiamano il diritto alla libertà di religione, compresa la libertà di convertirsi (non dimenticate che nei Paesi in cui vige la *Sharia* la libertà di convertirsi non c'è). Questo mi pare acquisito da tutte le forze politiche di questo Parlamento. Capisco che ognuno, se l'avesse scritto da solo, l'avrebbe fatto in modo diverso, ma questo è il bello della democrazia.

mi pare che la disputa di carattere semantico abbia risolto positivamente i dubbi residui sulla formulazione del documento, il quale, recando la firma di tutti i Capigruppo, non mi pare che abbia bisogno di ulteriori rifiniture o commenti. ragione, mi permetterei di sostenere l'opportunità di passare al voto dell'ordine del giorno senza bisogno di ulteriori dichiarazioni.

mi dispiace di non essere d'accordo su questo tema semantico con illustri colleghi, molto più esperti di me,

«Santissimo Padre», addirittura. Il concetto di santo sta a me a cuore, proprio perché venga definita la diversa autorità; non è una questione puramente ridicola. La parola «Pontefice» mi va bene se si scrive «Sua Santità Pontefice Massimo», ma non credo che andrà bene ad altri. Ecco la ragione per la quale insisto:

le ho dato la parola, ma questo documento ha una sua formalità: se confermato, è l'unico che oggi, dopo le dichiarazioni del Ministro, sarà posto in votazione.

disponibili ad adeguarci alla proposta del senatore Pisanu, con la raccomandazione però che le dichiarazioni di voto vengano consegnate alla Presidenza, se l'Aula è d'accordo.

semplicemente segnalare che, al di là dei problemi terminologici,

tratta di un'esigenza politica. Allora, se non possono essere svolte in quest'Aula, vi è una ragione di convenienza, per cui, quantomeno, devono essere formulate in forma scritta.

Grazie, mi pare che stiamo facendo il giro dei Capigruppo - così dovrebbe essere - perché si esprimano sulla proposta del presidente Pisanu. Non abbiamo difficoltà, ovviamente, a che si voti subito, ma chiediamo a tutti i colleghi - e credo che ciò sia nell'interesse di tutti i Gruppi - che si possano depositare, però, le dichiarazioni di voto, affinché parte integrante del resoconto, così come suggeriva il senatore Barbato. Mi permetto di svolgere due osservazioni. Innanzi tutto, desidero ringraziare il Ministro per l'attenzione con la quale ha seguito i nostri lavori e per il suo intervento, lucidissimo e colto, come sempre. Inoltre, desidero rivolgermi affettuosamente al presidente Selva. Presidente,

Glielo dico perché, appunto, considero questo un risultato non scontato in nessun modo. Mi consentano anche i colleghi - facendo una cosa che probabilmente sfugge a quello che è il protocollo ordinario fra di noi - di ringraziare, a nome mio personale e del mio Gruppo, la senatrice Albertina Soliani per il lavoro svolto in questi giorni, che ha consentito di arrivare al risultato di oggi. ringrazio, a nome della Lega Nord, per non aver aderito alla richiesta formulata da alcuni colleghi di rinunciare alle dichiarazioni di voto consegnando l'intervento. Ritengo che l'importanza dell'argomento dia diritto ai parlamentari che lo richiedano di esprimersi e, quindi, dopo le dichiarazioni di voto, di procedere al voto.

essa si è tenuta con grande rigore e serenamente. Il corteo è partito dal Colosseo ed è giunto a piazza Venezia. Qui accade qualcosa - e sono lieto che sia presente in Aula il Ministro dell'interno assolutamente intollerabile: non si consente a nessuno dei partecipanti al corteo di uscire dalla piazza. Si sta creando una situazione di enorme disagio. CORONELLA *(AN)*. *(AN)*. Il rigore con il quale si stanno trattando dei signori che legittimamente vogliono rassegnare alla pubblica opinione il loro disagio per questa situazione - che tutti noi conosciamo - complessa e dolorosa, per molti versi,

Signor Presidente, non voglio essere impopolare, ma visto che il Gruppo della Lega

sto soltanto dicendo che quest'atteggiamento va proprio nel senso dei discorsi che svolgiamo in quest'Aula. Uno dei maggiori obiettivi perseguiti costantemente dalla Chiesa cattolica, a cominciare da Papa Giovanni Paolo II, è stato quello di ispirarsi all'universalità e all'incontro fra tutte le religioni, la cui tendenza massima trascendentale è comunque quella di riferirsi a Dio,

ad un Dio di pace e non di guerra, di amore e non di odio, come ha testimoniato Cristo stesso e come professa lo stesso Islam. Questa apertura culturale, conclamata più volte con la *pellegrinatio* del precedente Pontefice verso altri Paesi ed altre culture, ha trovato punti di sublimazione nella richiesta di perdono in un anno significativo per tutta la cristianità come quello del Giubileo. Come non riportare la memoria, infatti, al 2000, che ha rappresentato un importantissimo traguardo sia per la Chiesa tutta, sia per lo stesso compianto Giovanni Paolo II, che ha traghettato con umiltà e devozione nel nuovo millennio un miliardo di cattolici, chiedendo umilmente perdono per gli sbagli commessi nei secoli dalla Chiesa, come ad esempio le crociate o l'uso di metodi non evangelici nel servizio della fede. è stata portata avanti da Benedetto XVI, se possibile, ancora con più calore. Ingiusto, quindi, è stato il frettoloso, probabilmente per alcuni strumentale, giudizio che, per le vicende che abbiamo appena ricordato, mai può attagliarsi alla figura di Benedetto XVI, le cui affermazioni, presso l'università di Ratisbona, sono state peraltro ispirate ad un dialogo fra l'imperatore Manuele II ed un saggio persiano, in un testo del lontano 1391! dialogo si estende su tutto l'ambito delle strutture di fede contenute nella Bibbia e nel Corano e si sofferma soprattutto sull'immagine di Dio e dell'uomo. Non possiamo poi non tener presente che i *media* non hanno citato per intero il periodo dal quale la frase contestata è stata estrapolata; in tal modo, non è stato pubblicizzato il contesto della stessa, aprendo così il campo a speculazioni e a reazioni ostili, specialmente di una parte del mondo musulmano, che ci hanno portato oggi Mai ci ha sfiorato il pensiero che il Papa avesse, con le sue parole, voluto in alcun modo offendere la sensibilità dei musulmani, poiché ben sappiamo come egli, al contrario, nutra verso la loro religione, come verso le altre religioni e culture, un atteggiamento di grande rispetto ma soprattutto di dialogo. Ciò che sta a cuore al Santo Padre, per suo stesso successivo, personale e sincero chiarimento, è un radicale rifiuto di ogni motivazione religiosa della violenza. Quindi, intristisce molto vedere come tutto il lavoro di apertura culturale, sin qui portato avanti con grande passione e trasporto dagli ultimi due Pontefici, possa essere, in modo anche un po' volgare, politicamente strumentalizzato. Ancor più intristisce apprendere che le parole di sincero rammarico del Papa non siano riuscite a placare le ire del mondo islamico più radicale, il quale ha sollevato una bufera che in, qualche modo, ha colpito le coscienze, la sensibilità e la vita di tutti noi. Queste vicende, per quanto stridano violentemente e nel profondo con le nostre radici culturali, non devono in alcun modo demotivare il Pontefice e tutti i cristiani nella ricerca di ciò che unisce, piuttosto di ciò che divide, poiché non deve mai essere dimenticato che, su questa terra, siamo tutti figli di un unico Dio. Altra cosa sono gli interessi particolari, le pulsioni umane non controllate dalla *ratio*, mentre le ragioni del trascendente ci unificano tutti inevitabilmente in un unico destino: polvere siamo e polvere ritorneremo. Laicamente bisogna tuttavia saper anche discernere. Chi vi parla è stato nel recente passato tra coloro i quali, in Campidoglio, hanno favorito l'edificazione ed il completamento della moschea, qui, nella nostra amata capitale, la capitale del cattolicesimo, come segno massimo di apertura e accoglienza. Devo sinceramente confessare che ripercorrerei senza indugio la stessa strada, ma vi accompagnerei una imprescindibile richiesta di reciprocità, come segno tangibile di comprensione dell'importanza di un gesto come quello allora da noi compiuto. La parità, la reciprocità, la volontà di approfondire la conoscenza della cultura e delle tradizioni altrui altrui denotano la profonda saggezza che vedo pervadere ed ispirare l'Islam moderato. Un esempio sicuramente lampante è proprio quello della vicina Turchia, ove persistono contemporaneamente frange, per fortuna minoritarie, di fondamentalismo accanto a classi dirigenti che sanno ben distinguere il laicismo di uno Stato libero e democratico dalla convinzione religiosa e l'estremismo strumentalizzato. Per tali motivi non posso che dimostrarmi ampiamente favorevole ad approfondire con serietà l'ipotesi dell'ingresso in Europa della Turchia. Sono, inoltre, assolutamente convinto dell'importanza altamente simbolica e culturale del viaggio di Benedetto XVI in quello stesso Paese e, sempre laicamente, chiedo che, per suggellare questa visita e per attribuirgli un significato di reale scambio culturale e di intelligente curiosità di conoscenza dell'altro, le autorità locali preposte, quelle turche, come accadde e accade già qui a Roma, favoriscano e si facciano promotrici di una rapida integrazione delle minoranze cristiane e cattoliche presenti sul territorio turco. Pertanto, daremo il nostro voto favorevole a tutte quelle iniziative, come questo ordine del giorno, che pongano come questione centrale ed imprescindibile il riconoscimento reciproco della libertà di religione e di cultura e la difesa dei valori, come quello della vita e del dialogo fra i popoli.

Presidente, mi parrebbe di sminuire l'importanza di questo tema ed anche il rispetto per la grande tensione della comunità, non solo di quella cristiana, se rinunciassi a una dichiarazione di voto. Mi sembrerebbe anche di sminuire il ruolo del Parlamento, che ha il compito di esprimersi su temi di grande rilevanza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la voglia di rivalsa, lo devo ricordare, errata e dannosa dopo gli attentati dell'11 settembre ha portato alla guerra dell'Iraq e ha alimentato lo scontro di culture e di religioni, uno scontro che tende a minacciare sempre di più la pace nel mondo e ci espone ad attentati terroristici. Abbiamo pertanto apprezzato il ruolo della Chiesa ed in particolare i messaggi commoventi di Papa Giovanni Paolo II in favore della pace, per il dialogo tra religioni e culture. Questa linea è stata pienamente proseguita da Papa Benedetto XVI, al quale vogliamo esprimere, a nome di tutto il Gruppo per le Autonomie, la nostra piena solidarietà. Respingiamo, pertanto, con fermezza le strumentalizzazioni della lezione sul rapporto tra ragione e fede tenuta dal Santo Padre all'università di Regensburg: era un'analisi storica che in alcun modo voleva essere di offesa al mondo islamico. Respingiamo quindi le minacce e gli attacchi ingiusti e inaccettabili rivolti al Papa e a tutta la Chiesa cattolica, attacchi e minacce mossi da una frangia, la più radicale, musulmana, ribelle, jihadista, antisemita e anticristiana, che si nutre purtroppo della disperazione di giovani emarginati e che ha come scopo quello di soffiare sul fuoco dell'intolleranza e della violenza. Il Pontefice, anche negli incontri con i rappresentanti islamici, ha ribadito invece la necessità di promuovere il dialogo interreligioso e interculturale fra cristiani e musulmani. Ha ragione il ministro Amato sul fatto che non dobbiamo scusarci per il discorso di Regensburg, ma dobbiamo ammettere naturalmente che anche la nostra religione, come tante altre nella loro storia, ha violato i propri principi etici. Noi, signor Presidente, crediamo che questa sia la strada giusta da seguire, assieme all'impegno che lo Stato deve mantenere nel contrastare fermamente ogni forma di violenza, di integralismo e di intolleranza. In tal senso, esprimiamo soddisfazione per l'azione finora svolta dal Governo e dalle forze di polizia. Questa azione deve proseguire a tutela del Pontefice, dei luoghi di culto e di tutti i cittadini. C'è bisogno di un dialogo autentico, che aiuti a superare insieme le tensioni, anche nell'incontro e nella convivenza con le comunità immigrate. Questo dialogo deve però prendere atto delle differenze e rispettarle, perché il rispetto reciproco è alla base di tutto e senza di questo non si può creare dialogo. Riteniamo, infatti, che siano importanti la libertà di religione, il rispetto dei valori ed anche la tolleranza, che per noi è un atto dovuto nell'incontro con le culture e le religioni di altri Paesi e nel confronto con le persone e le famiglie immigrate.

Chiediamo il rispetto del nostro credo, dei nostri simboli e dei nostri valori cristiani, che abbiamo il compito di sostenere. Vorrei essere molto esplicito su questo: non possiamo accettare che si chieda a noi di togliere la croce dalle aule scolastiche pubbliche, come noi non ci permetteremmo mai di chiedere questo ad altre religioni riguardo ai loro simboli nei loro Paesi. Puntando sul dialogo tra Paesi e popoli di culture e religioni diverse, fondato sulla parità, sulla reciprocità e sulla non violenza, si potrà scongiurare il pericolo di uno scontro tra le civiltà e le dignità culturali e religiose, quale unica deriva della crisi del nostro tempo. Pertanto, signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie

Provo un po' di imbarazzo, dopo avere ascoltato la discussione e anche rispetto all'ordine del giorno, che comunque il nostro Gruppo voterà, perché vi sono tre aspetti che secondo me dovrebbero essere chiariti e ben definiti, prima di procedere oltre. La prima questione, banale ma molto certa, è che non è compito di questo Parlamento fare l'analisi filologica o l'esegesi dei discorsi del Pontefice. E a parer mio non è compito di questo Parlamento nemmeno garantire sulle finalità e sulle intenzioni del Pontefice

e invece attestarci sul compito che questo Stato e questo Parlamento hanno di favorire la pace, il dialogo e le relazioni tra i popoli, tra le persone e gli Stati, in modo che questi non degenerino né in fanatismi, né in né in violenza né tanto meno in guerre. Devo anche dire, però, che sono rimasto abbastanza scioccato da alcune dichiarazioni e da alcuni peana sollevati dai Gruppi in quest'Aula. Ad esempio, quando sento il rappresentante della Lega Nord ergersi a strenuo difensore dei sacri valori del cristianesimo, e sicuramente interprete delle leggi divine,

che Dio perdoni! - portare la forca in Parlamento? Forse non ci capiamo su quali sono i valori cristiani e quale il valore della convivenza. convivenza. Anche in questo Parlamento tutti ci siamo espressi contro l'uso politico della religione e su questo sono d'accordo, come sono anche d'accordo sul fatto che meno si fa uso della religione

Quando poi sento la destra - non so se ancora si può chiamare così - dire che il grande problema è che le altre religioni non hanno un capo riconosciuto, non hanno la gerarchia, si tagliano 500 anni di dibattito, si taglia tutta la questione dei cristiani non cattolici. Forse perché la destra è così abituata alle gerarchie che, se non c'è una gerarchia, se non c'è qualcuno che deve sempre sottomettersi al volere altrui, non è in grado di recepire la libertà individuale, la sua irriducibilità, anche nel senso pieno della responsabilità. Probabilmente è questo il discorso. Di certo il problema del rapporto con le altre religioni che non hanno una gerarchia consolidata, come quella appunto della Santa Romana Cattolica Apostolica Ecclesia e del Servo dei servi di Dio, di Dio, mi pare davvero un'amenità storica e non degna di quest'Aula. Andando avanti su questo fronte, ho condiviso in parte le parole del Ministro dell'interno quando comunque fa l'autocritica; non ho condiviso il fatto che abbia detto «il nostro Dio», perché la Repubblica italiana non ha più una religione di Stato; è laica e garantisce le differenze etiche, le differenziazioni culturali e religiose a chiunque. a chiunque. Condividendo l'autocritica, fatta anche da altri onorevoli che sono intervenuti, devo però dire che questa certezza sul fatto che le religioni siano di per sé fattore di libertà, di emancipazione e di pace, e che questo sia poi il crisma della religione maggioritaria nell'Occidente, che, ripeto, non è solo il cattolicesimo, è il cristianesimo nelle sue differenti valenze, a me sembra un po' inopinata. Voglio ricordare solo l'ultima tragedia in cui non c'entra l'Islam: in Ruanda sono morte più di un milione di persone. Il Ruanda è un Paese al 90 per cento cattolico e al 10 per cento protestante. Vogliamo dire che anche quelli sono stati stati sollecitati dall'integralismo-fanatismo islamico o vogliamo forse capire che queste manifestazioni, o comunque questo uso delle religioni, è altro rispetto alla religione stessa? Quando sento dire, ad esempio, dall'ex ministro Buttiglione che l'Islam non ha compiuto il processo di liberazione dello Stato, e quindi di emancipazione della coscienza religiosa rispetto alla coscienza politica, posso essere anche in parte d'accordo. Tuttavia, vorrei ricordare che c'è un tentativo di cui Pera, ex presidente di questa Camera, si è fatto fortemente interprete: reintrodurre una battaglia contro il relativismo etico che - scusate - nella traduzione volgare di assolutismo etico, è nient'altro ciò che dice Mullah Omar, la teocrazia dell'Arabia Saudita e in parte anche alcuni teorici, secondo me anche poco avveduti, poco avveduti, del concetto di libertà dato da Dio rispetto alle proprie azioni e responsabilità. Ed allora di che cosa bisognava parlare e di cosa parliamo. Di una cosa giusta e necessaria ed è per questo che voteremo a favore della mozione. La cosa giusta e necessaria è il nostro rifiuto perché il dibattito perché il dibattito culturale e la contaminazione - perché vi è anche un sincretismo religioso - fra i vari credo, la possibilità di relazionarsi e di essere facitori di pace e di curiosità deve essere garantito contro violenze, intimidazioni

questo è il compito della nostra Repubblica e su questo crediamo molto. Devo anche dire che poco si è sentito sulla libertà di culto. Chi urla sulla libertà di religione non mi pare poi che nel concreto riconosca possibilità di culto alle altre religioni in questo Paese, se non rendendo difficilissima ogni opzione che non sia interna a quella della Sacra Romana Cattolica Apostolica Ecclesia. Concludo con un auspicio.

Anche Bush dice che Dio è con lui quando bombarda e i nostri cappellani militari ancora benedicono le armi come, credo, tutti i religiosi di tutto il mondo benedicono le armi dei loro Paesi perché lì è la volontà di Dio.

visto che la RAI ha preferito non far sapere come ben pensano, chi sono e come si comportano nei confronti di Sua Santità

Non dobbiamo dimenticare che i nostri martiri - la nostra gente - muoiono per un progetto di amore, mentre i martiri per l'Islam muoiono

Il Primo ministro, però, come cittadino e cristiano cattolico mi ha lasciato fortemente perplesso e preoccupato. È proprio su questo punto che voglio spendere i miei pochi minuti di intervento, pervenendo ad una riflessione che voglio svolgere ad ad alta voce. È risaputo che il progetto massonico teorizza che il modo migliore per controllare socialmente demograficamente l'umanità è la diffusione del vizio e dell'immoralità e la creazione di società multirazziali, con lo scopo preciso - c'è, infatti, uno scopo preciso - di rovesciare e distruggere il cristianesimo, unico punto di forza e testimone fondante della nostra società. Non faccio il poliziotto di mestiere, ma mi riferiscono che il nostro Presidente del Consiglio è un frequentatore assiduo di logge massoniche che in una *convention* ad Aquisgrana, negli anni Ottanta, è stato investito di grande poteri e responsabilità.

il disinteresse di una civiltà che il nostro Presidente - se questo mondo serve - spero vorrà abbattere. La logica l'ho trovata nel cognome del nostro Presidente del Consiglio:

è diventato un soldato di Cristo e come tale non può delegare ad altri la sicurezza del Santo Padre;

Penso che il nostro compito sia quello di attivarci in tutti i modi per garantire a Benedetto XVI una lunga vita perché con i suoi insegnamenti possa illuminare le nostre menti oscurate in un momento di secolarizzazione della nostra società.

Cosa dire poi del rifiuto dell'Europa nell'inserire nella propria Carta costituzionale le radici cristiane? Il nome Benedetto, scelto dal cardinale Ratzinger è un messaggio preciso al popolo cristiano, perché San Benedetto fu il primo a raccogliere i resti dell'impero romano e a organizzare territorialmente la nascita di un'Europa con le fondamenta cristiane fino in fondo.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il dibattito nato con le dichiarazioni di voto ha messo in evidenza quanto la scelta che stiamo compiendo sia importante e anche difficile.

dichiarino di essere uniti nel sostegno all'azione di pace e di dialogo fra religioni e anche di dialogo nella verità iniziata da Benedetto XVI. Perché il dialogo chiede identità, altrimenti non è dialogo, ma è cedimento. Benedetto XVI è entrato in questo dialogo con una identità forte che, io credo, non è soltanto l'identità dei cristiani, ma è l'identità dell'Occidente: un'idea di libertà, un'idea di verità e un'idea di ragione. Vi è entrato anche con una critica del nostro Occidente. Vorrei dire al ministro Amato, che però non vedo, che nell'intervento del Papa c'è la piena comprensione della fatica che l'Occidente ha fatto per costruire questa idea di verità, a partire da una inevitabile base cristiana. Crediamo noi che l'Islam possa evolvere in questo senso? Certo che lo crediamo. Crediamo che l'Islam oggi ci sia? Ancora non c'è, tanto è vero che è scisso ed esistono delle tendenze integralistiche che sono un'effettiva minaccia. Vorrei dire che se aprissimo un dibattito culturale, vi sarebbero molte cose su cui dissento dal ministro Amato. Quanto a questa idea del risentimento del mondo arabo contro il colonialismo occidentale, lo sa il ministro Amato che l'Arabia Saudita non è mai stata

anche perché le crociate furono la risposta alla *Jihad*, alla guerra santa, che aveva occupato territori precedentemente cristiani. Capisco la difficoltà che ha il ministro Amato nel tenere assieme una maggioranza la quale ha opinioni molto diverse su questi temi,

negli anni Trenta, con il movimento di liberazione arabo che poi si concretizza nel partito Baath, che guarda con grande ammirazione all'Italia, a Benito Mussolini, alla Germania, ad Adolf Hitler. Non dimentichiamo queste radici vere, concrete. *(Applausi dai laico fallisce - e fallì con Nasser - allora Said Qutb inizia a tradurlo in termini religiosi. L'integralismo islamico ha poco a che fare con la storia millenaria dell'Islam, o, meglio: ha a che fare con la storia millenaria dell'Islam, ma ha a che fare anche con questo nazionalismo esagerato che si ritraduce in termini fascisti e nazisti. Quando si parla di fascismo islamico, di nazismo islamico, non si hanno tutti torti. Davanti a questo è giusto che ci difendiamo perché siamo gli aggrediti. Non dimentichiamo che è sempre bene bene avere memoria del passato, ma è anche bene avere memoria corretta del passato e affrontare i problemi del presente. Detto questo, voterò a favore di questa mozione che rappresenta un momento alto di convergenza di diversi nell'affermare alcuni valori irrinunciabili, costitutivi dell'identità del popolo italiano.

suscita in me vera gioia, grande compiacimento, constatare tanto spirito solidale e filiale dell'Aula verso il Santo Padre. Un Santo Padre che anch'io amo, quale capo della spiritualità cristiano-cattolica; che amo con la consapevolezza, pari al rammarico, di non essere costantemente e in ogni situazione degno, secondo aspettativa, del Padre dei Padri di tutti e di ciascuno di noi, credenti, non credenti, atei, agnostici.

che non ho sottoscritto la mozione, depositata dal mio Gruppo parlamentare di appartenenza agli atti di questo ramo parlamentare; non l'ho sottoscritto in quanto persuaso che non tale documento, ma ogni e qualsiasi documento analogo, quindi anche quello compilato dai Capigruppo, manifesti profili di lesività del principio di sovranità democratica del Parlamento. Un principio, quello della sovranità democratica, che non può contemplare più tipi di attori, uno solo, il cittadino, essendo la ragione d'essere stessa della sovranità democratica. Ma un cittadino, quello che sta nella mia preferenza, che vive la propria fede come un libero impegno della sua coscienza, non già, giammai, come un credente che più o meno in buona fede, in nome della volontà di Dio magari, indulge in pressioni per sospingere in avanti la propria religione. Com'è chiaro,

Una laicità da non vedersi come pura e semplice separazione e neutralità in tema di confessioni religiose, quanto e unicamente quale condizione per la realizzazione di una vera Città politica. Una Città che tutto comprenda, come nel nostro Paese tutto comprende. Anche Chiesa e culti religiosi, in posizione rilevante e significativamente positiva. Una laicità che seguendo il tracciato del pensiero cartesiano è sinonimo di generosità, in quanto accredita a ogni essere umano la libertà e la facoltà di servirsene bene, come scriveva recentemente il noto filosofo contemporaneo Henri Peña-Ruiz. Ma badate, signori senatori, la generosità laica, soprattutto quella laica dell'uomo di fede, è rifiuto del paternalismo ed invece è premessa che unisce gli esseri umani e li accomuna al di sopra dei loro particolarismi. E qui, a questo punto, come non dire che siamo al centro del centro del messaggio religioso-esistenziale del Concilio Vaticano II? Ma se così se così è, la generosità laica di ciascuno di noi verso il Santo Padre a me pare debba consistere anche nell'avere la temperanza, la saggezza di non parlare al guidatore. Riconoscendo che ciò di cui Egli ha bisogno è il conforto della preghiera incessante dei credenti, non meno della fiducia e del calore dei non credenti e degli atei in ordine al suo essere valore universale di bene e di amore per l'uomo. Da laici, non perdiamo la memoria storica. Ricordiamoci che le contiguità e i collateralismi fra potere politico e potere religioso, sempre e sistematicamente sono stati nefasti. sono stati nefasti. Spesso sono sfociati in derive clericali. Così dall'imperatore Teodosio (380 d.C.); così dal fenomeno dell'*Ancien Régime*; così dal Syllabus; così dalla collusione di Papa Ratti con il fascismo. Penso, amici del Senato, di aver espresso lievemente e come si può in poco tempo,

per una ragione politica sostanziale: abbiamo così voluto contribuire ad una non divisione di questo ramo del Parlamento su una questione di tale delicatezza e complessità. Allo stesso tempo però, e proprio questo dibattito per certi versi così pacato e civile lo conferma, stiamo parlando di questioni così complesse e difficili che la politica - sottolineo: la politica, non questo ramo del Parlamento - ha una grande difficoltà a rappresentare la molteplicità delle sensibilità, delle culture e dei punti di vista individuali. Questa difficoltà di rappresentazione ci ha spinto dunque a considerare, per il nostro Gruppo e per i nostri senatori, la libertà di voto e anche di non voto. Colgo l'occasione di questa circostanza per esprimere un forte apprezzamento per il contributo

ispirato ad uno dei cardini della nostra visione di questi problemi, ovvero il rovesciamento - ne parlerò meglio tra qualche minuto - della tendenza più pericolosa in atto nelle nostre società,

tale si può chiamare, che si è svolto oggi in Parlamento è funzionale anche a questa visione. Vorrei richiamare brevemente le due questioni principali che sono state oggetto delle riflessioni e degli interventi.

Mi pare ormai sia chiaro a tutti che ogni interpretazione strumentale, fanatizzante o tendente addirittura all'assunzione di una sorta di nuova guerra di religione sia da considerarsi infondata. Il Pontefice ha dato prova di notevole saggezza politica e di notevole abilità diplomatica, pur esprimendo certo una visione culturalmente molto definita. Credo che, al di là dei grandi problemi irrisolti che si pongono sullo sfondo di quella lezione, delle reazioni e delle minacce che essa ha suscitato, dovremmo considerare chiuso non l'incidente, ma la propensione che ogni tanto è comparsa e che ogni tanto ricomparirà a tirare il Pontefice per la giacca, anzi - come sarebbe più appropriato dire - per la tonaca. Penso ci sia qualcosa di irrispettoso, forse persino di dissacrante, in questa tentazione di utilizzare le parole del Pontefice, del capo della cattolicità, per fini di parte o di propaganda politica.

la morale cattolica come fonte di legittimazione della morale pubblica e, addirittura, della legislazione italiana,

analitico rilevante anche per il nostro comportamento, le nostre scelte e le nostre battaglie. La seconda questione su cui volevo soffermarmi ha ha costituito l'oggetto centrale dell'intervento di Giuliano Amato: è il pericolo dello scontro di civiltà che incombe sulle nostre società. Non abbiamo il tempo per un'analisi approfondita che sarebbe certamente necessaria. Voglio solo sottolineare che tale questione, in particolare dall'11 settembre 2001 in poi, si sta esprimendo non solo nella tragica spirale guerra‑terrorismo che attanaglia il pianeta, ma in una crisi più profonda della stessa civiltà occidentale, dove sono finite le grandi narrazioni novecentesche e dove rischiano di smarrirsi certezze e valori condivisi, talora perfino il senso della vita. La pianta del fondamentalismo cresce in questo quadro e in questa crisi: è una risposta semplificata e fanatica, una scorciatoia identitaria e un elemento inquinante che contiene in sé violenza morale e materiale. Quando dico fondamentalismo - lo voglio sottolineare - aggiungo anche, però, che non è esatto identificarlo con islamismo, come si tende impropriamente a fare. Il fondamentalismo è in crescita in tutte le religioni e in tutte le culture. C'è anche, per esempio, il fondamentalismo del mercato che fa della sua logica l'unica possibilità di salvezza per le società. C'è il fondamentalismo laicista, c'è perfino un fondamentalismo della scienza e dell'Occidente come

necessità e dell'urgenza di contrastare tale tendenza, di marginalizzarla e combatterla culturalmente, a partire, appunto, dalla parola d'ordine del dialogo delle civiltà. Non lo facciamo solo in nome degli antichi valori europei di cui siamo portatori e eredi orgogliosi, come il dialogo, il confronto e la custodia dei valori di libertà; lo facciamo anche in nome dei valori nuovi

del meticciato, della contaminazione e dell'incontro, di una crescita dell'umanità e delle culture che può avvenire oggi in un mondo sempre più grande grande e incontrollabile, ma sotto molti aspetti sempre più piccolo. Può avvenire qualcosa che non è mai avvenuto finora. Lo ripeto:

«nuova identità umana», rispetto al quale le battaglie, anche della sinistra, oggi possono collocarsi, attraverso l'assunzione dell'ottica, della teoria e della pratica della non violenza. Ho concluso, signor Presidente, e spero di non avere debordato oltre il tema che ci era prospettato.

Signor Presidente, signor Ministro - che non vedo -, colleghe e colleghi, quella che stiamo svolgendo non è, né può essere, una discussione di carattere teologico. Come ben ricordava il senatore Buttiglione, non può essere neanche l'occasione per revisioni storiografiche. Al Ministro dell'interno vorrei dire che, se ne ha voglia, ci sono sedi diverse per approfondire la questione delle crociate o l'esegesi di locuzioni evangeliche. Vorrei solo aggiungere in relazione al suo discorso - che mi sembra scritto più con il compasso che con la penna - *(Applausi dai nell'VIII secolo, a Lepanto sul 1571, sotto le mura di Vienna nel 1683 non è qualcosa di cui vergognarsi, ma è qualcosa di cui essere fieri come occidentali;

Se oggi non siamo un Paese islamico e se oggi tante colleghe contribuiscono in modo felice e determinante ai lavori anche di questo Senato invece di essere costrette a casa sotto un *burqa*, lo si deve anche al sacrificio degli eroi di Poitiers, di Lepanto e di Vienna. Non possiamo e non dobbiamo esprimere valutazioni sulla lezione del Santo Padre a Regensburg, non ci compete. Questo voto non è né pro né contro il Pontefice; Pontefice; il suo tema centrale - che è anche l'oggetto principale dalla mozione - è quello della libertà religiosa. Su questo vorrei spendere qualche parola perché sul tema delicato dei rapporti tra religione, cultura e politica il dibattito pubblico sembra quasi bloccato. Sembra che esistano solo due posizioni: da un lato il laicismo e dall'altro il fondamentalismo, quando invece le opzioni sono quantomeno tre. Vi è certamente l'opzione laicista del potere tecnico fine a sé stesso, per la quale conta esclusivamente il *know-how* e la religione è ridotta ad una dimensione esclusivamente privatistica, sicché tra fede, cultura e politica esiste un muro invalicabile. Vi è, certamente, l'opzione fondamentalista, tipica oggi del radicalismo islamico, per la quale religione, cultura e politica coincidono. Vi è, tuttavia, una terza ipotesi, quella che non conosce una separazione netta e radicale tra fede, cultura e politica, ma riconosce loro una opportuna distinzione. Si tratta di quella che è stata chiamata la laicità positiva, per la quale ci sono princìpi di diritto naturale riconoscibili da chiunque sui quali si fonda il nostro vivere civile, ma che sono negati sia dal fondamentalismo laicista, sia da quello di altre confessioni religiose. Questi diritti sono riconoscibili con l'uso di ragione e in questo la nostra cultura differisce dal radicalismo islamico. Tali diritti includono quello a professare liberamente la propria fede; includono, cioè, la libertà religiosa. Quando in Stati con i quali abbiamo intensi scambi economici e commerciali la fede diventa elemento di discriminazione e di persecuzione, il tema acquista una drammatica concretezza e perde ogni connotato di astrattezza. Dovremmo disinteressarci, come ha fatto il Presidente del Consiglio nel suo recente viaggio in Cina, della sorte di migliaia di fedeli cinesi di svariate confessioni religiose: dai protestanti ai musulmani, dai buddisti ai tibetani, dal Falun Gong fino ai cattolici? Dovremmo ignorare, sullo stile del presidente Prodi, la lista interminabile di vescovi e di sacerdoti, talora ultraottantenni, arrestati, detenuti, torturati o comunque impediti nel loro ministero? La lettura dei nomi dei religiosi che solo in Cina sono stati fatti scomparire senza lasciare tracce farebbe superare abbondantemente i dieci minuti oggi a mia disposizione. Non parlo ovviamente di ciò che accade nei Paesi a maggioranza musulmana perché è troppo noto e le condanne a morte delle ultime settimane lo confermano. Comunque, non è necessario andare così lontano perché quando un altro Parlamento, come quello europeo, considera ostativa per l'incarico di Commissario europeo un'opinione frutto di un'impostazione etica ed, in ultima analisi, religiosa - è il caso del collega Buttiglione vuol dire che c'è qualcosa di cui preoccuparsi anche dalle nostre parti! (*Applausi dai Gruppi AN, UDC e FI)*. Ciò può apparire paradossale, ma è significativo. Radicalismo islamico e fondamentalismo laicista convergono nel perseguire i medesimi risultati di marginalizzazione della religione dalla nostra vita quotidiana. Sul rifiuto del riconoscimento della libertà religiosa si fonda la reazione irrazionale e fanatica alle parole del Santo Padre a Regensburg: si fonda cioè sull'irrazionale rifiuto di constatare che la religione non ha soltanto

si vuole impegnare il Governo a rendersi promotore nelle istituzioni europee di iniziative che tutelino la libertà religiosa. Siamo lieti che il Senato nella sua interezza voti questo importante documento; siamo lieti che ciò avvenga su iniziativa delle forze politiche della Casa delle libertà. Abbiamo soltanto il rammarico di non averlo potuto fare tempestivamente, visto che qualche settimana fa, nell'imminenza dei fatti gravi, il Senato con un solo voto di scarto ci ha impedito la possibilità di discuterlo. Non è mai, però, troppo tardi! giorno si vuole impegnare il Governo ad impedire che il richiamo religioso sia strumentalizzato per atti di violenza o di intimidazione: deve farlo, però, non in modo generico o astratto, ma con misure concrete; farlo, signor Presidente, senza condividere la formula attribuita di recente al primo ministro spagnolo José Luis Rodrìguez Zapatero, secondo cui oggi la religione è il tabacco del popolo. di una formula che fa pensare, perché in qualche misura aggiorna l'espressione "oppio del popolo". Mentre l'equivalenza marxista tra religione ed oppio riflette ancora un approccio violento il tabacco evoca invece un tratto a metà tra il divieto e la tolleranza: il tabacco è escluso da qualsiasi spazio pubblico, scuole, parlamenti e luoghi di lavoro; se proprio qualcuno si ostina a voler accendere la sigaretta deve farlo in luoghi appartati, deve stare a distanza dal suo prossimo, deve evitare la propalazione del fumo passivo, deve portare in giro pacchetti pieni di scritte contro il fumo. Se è valida l'analogia, sostituite al tabacco la religione intesa in senso ampio. Nell'accezione laicista va trattata alla stessa maniera: la religione - e più in generale ogni discorso relativo a princìpi o a richiami etici - andrebbe tenuta a distanza dai luoghi pubblici, andrebbe etichettata come gravemente nociva alla salute, ne andrebbe vietata la propaganda soprattutto ai minori

di eredi di una tradizione che anche per chi non crede è una tradizione cristiana, impedire che la cosiddetta legge Sirchia sia estesa alla religione e a quei princìpi per i quali vale la pena di lottare e di impostare anche l'impegno politico.

Signor Presidente, comprendo che le conclusioni di questo dibattito, che giudico molto positive, abbiano fatto venire più di qualche mal di pancia ad alcuni colleghi senatori; per questo vi è stato il tentativo di gettarla chi in accademia, chi in sagrestia, chi infine perfino in goliardia. Ma vorrei che noi stessimo al punto politico di questo dibattito, quello che evidentemente più ci compete.

Su questo concordo con la collega Brisca Menapace: ne avremmo potuto fare a meno, se non altro per motivi di stile. Chiunque conosca i canoni della retorica medievale ai quali quel discorso si rifà, sa che Benedetto XVI non aveva fatto sue le parole del imperatore bizantino, dalle quali il suo discorso aveva solamente retoricamente preso le mosse. Ma non è questo il punto. Il punto è un altro: e se anche le avesse condivise quelle parole? *(Applausi dal Gruppo FI).* Avremmo potuto ritenere inopportuno il suo comportamento, lo avremmo potuto criticare dal punto di vista diplomatico, ma mai avremmo dovuto ritenerlo responsabile delle violenze che il suo discorso ha scatenato e che hanno portato alla morte di Suor Lionella alla distruzione di alcune chiese. Questo è il vero punto politico. Questo episodio, si dirà, si inserisce nel quadro di un più lungo attacco nei confronti della cristianità e dell'Occidente, che in particolare si è acuito dopo l'11 settembre 2001.

del ministro Amato. Nell'ascoltare il suo invito a storicizzare e i suoi richiami alla responsabilità del colonialismo occidentale

non hanno alcun tipo di sostanza e fondamento. Il problema sarebbe piuttosto indagare cosa è successo nel mondo islamico dagli anni Ottanta ad oggi e come

ministro Amato, piuttosto che richiamare la condizione delle donne islamiche che vivono segregate nel nostro Paese - e la pregherei di considerarle anche nel momento in cui c'è da discutere di immigrazione, essendo un po' meno meno lascivo nei confronti degli schemi del multiculturalismo che costringono quelle donne a una condizione di segregazione *(applausi dal Gruppo FI)*, perché riconoscono i diritti della comunità

di ogni atteggiamento che lede la possibilità di esprimersi. Credo che in questo emiciclo molti colleghi, anche dell'altra parte, si siano accorti che non a caso, dopo il discorso di Ratisbona, è stato censurato Mozart si siano chiesti, come me, quando verrà censurato Dante e verranno posti i puntini sospensivi in luogo di alcune espressioni usate dal sommo poeta. *(Applausi

Vuole invece essere un aiuto concreto ai tanti cristiani che si trovano a testimoniare il loro impegno in zone difficili del mondo,

che, per il consenso unanime del Senato, costituisce il segno di una nuova fondata speranza, che è un impegno forte dell'Italia. Il Gruppo dell'Ulivo è lieto di avere dato forza a questa speranza e a questo impegno. Signor Presidente, considerate le circostanze temporali, poiché penso che le parole impegnative abbiano bisogno di un contesto impegnativo e, soprattutto, poiché è più importante il voto che insieme ci apprestiamo ad esprimere, lascio agli atti la mia dichiarazione di voto, non senza aver fatto notare che l'ordine del giorno è firmato da tutti i Capigruppo del Senato della Repubblica in ordine alfabetico. Non so se sia la prima volta, certo è un segno nuovo nella politica italiana: insieme, alla pari, con l'umiltà, il rispetto, la misura che le cose grandi che ci sono di fronte richiedono. Oggi, signor Presidente e cari colleghi, è una buona giornata. Grazie.

L'ordine del giorno li ha fugati, ma una parte del dibattito li ha confermati. Desidero perciò sottolineare che darò il mio voto favorevole considerandomi del tutto estraneo a qualsiasi tentativo di strumentalizzare i valori religiosi a fini politici, perché questa è la cifra di tutti i fondamentalismi che impestano il mondo.

L'onorevole Soliani ha attribuito un qualche valore all'ordine alfabetico; a maggior ragione potrei io attribuire un valore politico al significato dell'attribuzione

quando valori che attengono al grande messaggio del Pontefice romano saranno da tradurre in pratica. Quella sarà la prova concreta di un'unità vera

Se le ho capite bene, esse possono riguardare tutti e ciascuno di noi. Ho ascoltato con una certa sofferenza interventi che davano per scontato premesse, culturali ed ideologiche, sulle quali mai potrei consentire.

che quando sento parlare di miseria dello storicismo mi vengono i brividi. Ma non è questa la sede per rivendicare l'altezza, la grandezza di un pensiero che ha fatto la cultura contemporanea e anche la nostra cultura di italiani

L'impegno dei Capigruppo e di coloro che hanno lavorato a stretto contatto con loro ha prodotto un testo laicamente condivisibile da molti di noi, e forse da ciascuno di noi. Si tratta, tuttavia, di un testo che il Senato vara qui, su cui esprime un voto, che non vincola il nostro pensiero, le nostre opzioni, la nostra libertà di essere credenti e non credenti, perché altrimenti si stabilisce un precedente

ma desidero sia precisata l'interpretazione che ritengo si debba dare all'ottica della reciprocità che compare nell'ultimo paragrafo del testo. Il principio di reciprocità implica un criterio di scambio e io non credo che il problema della libertà

Signor Presidente, intervengo per fatto personale personale poiché un collega, precedentemente, nel suo intervento in dichiarazione di voto sull'argomento oggi all'ordine del giorno, non so per quale motivo - forse non lo sa nemmeno lui, perché si tratta ovviamente di ignoranza nella materia politica in senso generale - ha confuso il simbolo di un partito con la sua critica e ha voluto nominare un collega oggi assente, il segretario di un partito che non ha il simbolo che lui ha denunciato, volendolo strumentalizzare per una sua opinione,

un argomento che è già stato toccato questa mattina dal collega Valentino. Avendone, peraltro, signor Presidente, avuto cognizione diretta e avendolo sperimentato sulla mia persona, come su quella dei colleghi Giuseppe Menardi e Andrea Pastore, credo sia necessario denunciare all'Assemblea che cosa è accaduto questa mattina nel cuore di Roma. Abbiamo assistito, signor Presidente, alla prima prova, riuscita, di un autentico Stato di polizia. Il cuore di Roma, a fronte di una manifestazione assolutamente pacifica, che non dava motivo alcuno di preoccupazione per ciò che atteneva all'ordine pubblico, è stato letteralmente sigillato, impedendo ai cittadini di transitare, addirittura laddove vi fossero le più elementari esigenze da soddisfare. I parlamentari sono riusciti a transitare attraverso piazza Venezia solo dopo ripetute insistenze. Cordoni tripli di Polizia e Carabinieri, automezzi che sigillavano completamente ogni varco e questo solo, signor Presidente, perché questa mattina vi era una manifestazione di professionisti che in alcun modo dava preoccupazioni di sorta. Mi chiedo, signor Presidente, memore anche di ciò a cui abbiamo assistito nei cinque anni precedenti, quando liberamente si veniva a manifestare sotto il Senato della Repubblica e sotto la Camera dei deputati, cosa sarebbe accaduto. Oggi abbiamo assistito a persone anziane a cui è stato impedito di raggiungere un bar, sequestrandoli di fatto da una parte all'altra di piazza Venezia. Riecheggiano, allora, le parole del Presidente del Consiglio, quando ha cupamente minacciato coloro che avessero avuto l'ardire di scendere in piazza. Stamani abbiamo capito per la prima volta cosa volesse dire. La nostra voce, signor Presidente, non la farà tacere nessuno. Risuona oggi qui, risuonerà alla Camera e faremo in modo che continui a risuonare nel Paese.

Signor Presidente, sono costretto ad intervenire brevemente per una puntualizzazione rispetto a quanto accaduto ieri in Aula, durante la votazione pomeridiana. A differenza di quanto riporta la stampa odierna, che vorrebbe far pensare ad una mia assenza volontaria dall'Aula, unitamente al senatore Formisano, al momento della votazione delle dimissioni della senatrice Turco, rispondente, chissà, a quale fantomatico disegno politico, voglio precisare semplicemente che la mancata presenza alla suddetta votazione è derivata da un semplice allontanamento dall'Aula, nell'errata considerazione che la votazione si sarebbe svolta